Signor Presidente, mi auguro che in Aula regni la dovuta attenzione rispetto a questo argomento. Le chiedo di richiamare i colleghi, grazie. per cortesia un attimo di attenzione: la senatrice Rauti sta illustrando la mozione n. 49 che credo interessi a tutta l'Assemblea.

che quest'Assemblea voglia compiere un gesto importante sottoscrivendo con un consenso trasversale tutte le mozioni presentate. nostra mozione la settimana scorsa, in vista di una scadenza, quella del 25 novembre, data in cui ricorre la Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne istituita, com'è noto, dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite nel 1999. Tale istituzione invita i Governi, le organizzazioni internazionali e le organizzazioni non governative a intraprendere iniziative di sensibilizzazione dell'opinione pubblica sul tema della violenza di genere. La Giornata, chiaramente, rientra in un perimetro internazionale molto solido su questo tema. Vent'anni prima della sua istituzione, l'Assemblea delle Nazioni Unite ha adottato la convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti delle donne. E ancora, voglio ricordare - perché resta un punto di riferimento ineludibile - la quarta conferenza mondiale delle Nazioni Unite che si è svolta a Pechino nel 1995, che stabilì in maniera definitiva che i diritti delle donne sono diritti umani e che le violenze di genere sono una violazione dei diritti umani fondamentali. Evidentemente, poi, il perimetro si rafforza con molte convenzioni con molti accordi internazionali ed è doveroso citare fra queste la Convenzione di Istanbul, approvata nel 2011, che introduce sulla materia,

tutta la Convenzione sostanzialmente a tre princìpi: quelli di prevenire il fenomeno della violenza, di proteggere le vittime della violenza e di punire gli autori della violenza. Nonostante vi sia un perimetro internazionale di riferimento forte e una normativa italiana solida su questo versante, su questo fronte (e potrei dire su questa trincea), l'Organizzazione mondiale della sanità continua a ricordarci ogni anno, cifre e stime alla mano, che la violenza di genere è una questione strutturale, un fenomeno di dimensioni globali, un mondo che attraversa il mondo, una questione trasversale alle religioni, alle geografie ai ceti sociali, alle appartenenze di società, quindi qualcosa di veramente e drammaticamente più profondo. Purtroppo ogni anno, anche in questo Paese, si continuano a registrare atti di violenza sulle donne e i cosiddetti femminicidi, ovvero quegli omicidi di donne basati su una basati su una motivazione di genere, ovvero l'uccisione di una donna in quanto donna. L'Eures ci ricorda addirittura che ogni due giorni e mezzo, ogni sessanta ore, una donna viene uccisa in ragione del suo essere donna e quest'anno già abbiamo dovuto, purtroppo, tenere il macabro conteggio di 65 vittime e la cronaca ci continua ad offrire ogni giorno casi di violenza e ogni due giorni e mezzo casi di femminicidio. L'Italia ha fatto molto in termini normativi, ma ancora resta qualcosa da fare. L'Italia è intervenuta, forse con un certo ritardo rispetto agli altri Paesi europei, con la prima legge organica del 1996, che per il nostro Paese costituì uno spartiacque fondamentale, un punto, per fortuna, di non ritorno, perché quella legge stabilì una volta per tutte che i reati di violenza non erano reati contro la moralità pubblica e il cosiddetto buon costume, ma erano finalmente riconosciuti come reati contro la persona. Un altro tassello normativo importante è sicuramente rappresentato dalla legge del 2009, più nota come cosiddetta legge anti-*stalking*, che andava a colmare un vuoto normativo e a punire quelle condotte reiterate e ripetute di molestie nella loro vasta gamma. E ancora, un altro pilastro è rappresentato dalla legge n. 119 del 2013. Noi abbiamo rivolto al Governo questa mozione chiedendo alcuni impegni, taluni dei quali ho visto che ricorrono anche nelle mozioni che sono state presentate dopo la nostra. Evidentemente indichiamo tutti un bisogno, anche perché nel contratto di Governo non c'è su questa materia una parte esplicita e allora noi chiediamo al Governo degli impegni precisi, a cominciare dalla piena attuazione del Piano nazionale antiviolenza previsto dalla succitata legge, ovvero la n. 119 del 2013. E ancora, chiediamo al Governo di intraprendere tutte le opportune iniziative di competenza al fine di garantire la protezione delle donne e dei loro figli e su questo anticipo che stiamo lavorando ad interventi normativi che non potevano trovare posto, evidentemente, in una mozione.

a garantire che le risorse ripartite nella Conferenza Stato-Regioni (a cominciare da quelle stanziate nella Conferenza del maggio 2018) siano erogate sempre, con regolarità

cosiddetti orfani di femminicidio (ossia gli orfani di crimini domestici), al fine di renderla pienamente operativa. Si chiede altresì di informare il Parlamento sulle attività della cabina di regia prevista per dare impulso alle politiche in oggetto, nonché su quelle svolte dal neonato Comitato tecnico

che tutti i colleghi sappiano che Fratelli d'Italia ha aderito a una campagna, che è diventata trasversale, intitolata: «Non è normale che sia normale», che ci siano omicidi di donne, violenze domestiche e stupri. Non è normale abituarsi a questo e non ci vogliamo rassegnare, perché rassegnarsi significa rendere normale ciò che - invece - è mostruoso. In conclusione, desidero fare una citazione. In genere, a margine di

che invito i colleghi e le colleghe ad ascoltare: «Per tutte le violenze consumate su di lei, per tutte le umiliazioni che ha subìto, per il suo corpo che avete sfruttato, per la sua intelligenza che avete calpestato, per l'ignoranza in cui l'avete lasciata, per la libertà che le avete negato, per la bocca che le avete tappato, per le sue ali che avete tagliato, per tutto questo: in piedi, signori, davanti ad una Donna».

Uso la parola civiltà non a caso, perché ha a che fare con l'idea di società che abbiamo in mente: una società aperta o una società chiusa in cui si tutelano e si difendono, forse anche per inerzia e pigrizia mentale, i tabù del passato e gli stereotipi per cui, quando si parla di violenza contro le donne si ha in mente soltanto la violenza sessuale. In realtà è qualcosa di più, forse di più sottile, di più profondo, di più pericoloso, che mette insieme le molestie fisiche

limitata. Molto spesso percepisco, anche in quest'Aula, un fastidio nei confronti dell'estensione dei diritti civili, quando invece l'avanzamento dei diritti civili e politici, insieme a quelli economici e sociali, ha garantito la crescita delle nostre società. Questo è un punto fondamentale. È una battaglia in cui non possiamo lasciare le donne da sole: è una battaglia che tutti insieme, uomini e donne, dobbiamo portare avanti. Lo dico soprattutto guardando i numeri, che sono riportati nella nostra mozione, che fanno solo immaginare la portata, la dimensione e la gravità di questo fenomeno.

la violenza viene dall'ambito familiare, quello in cui ci si fida di più e si abbassano le difese. Questo fa pensare che siamo di fronte ad un'emergenza nel nostro Paese, che non può essere sottovalutata. Nella precedente legislatura si è fatto un passo in avanti notevole, grazie ai Governi Letta, Renzi e Gentiloni ricordare l'atto più importante, quello che ci ha visto ratificare insieme la Convenzione di Istanbul nell'ambito del Consiglio d'Europa: parto da questo primo strumento internazionale vincolante

come il Consiglio d'Europa. Tuttavia, è proprio grazie alle organizzazioni sovranazionali che abbiamo fatto un passo in avanti notevole nell'estensione dei diritti civili e politici

per la prima volta il tema di essere liberi dalla violenza viene scritto in un atto europeo. Non è una concessione, ma un diritto e il tema della parità di genere è strettamente correlato e legato a quello della violenza. Quindi, se agiamo sul tema della parità di genere, creiamo una società più aperta e più libera, in cui finalmente si in qualche modo affermare quelle libertà che possono sfondare il soffitto di cristallo che ancora tarpa le ali ai talenti femminili.

il lavoro fatto nella sanità, con le corsie preferenziali per le donne che hanno subìto violenza; il lavoro nell'ambito della magistratura, con le nuove linee guida del Apro una parentesi, ricordando al ministro Salvini, che ieri parlava della grande innovazione del codice rosso, che esso si trova già nella legge sul femminicidio, portata avanti

Completiamo il lavoro sulla Convenzione di Istanbul, a partire dall'articolo 17, sulla comunicazione. Esso investe i *media* e il modo e il linguaggio che mettiamo in campo per raccontare la violenza contro le donne. Attenzione a non usare espressioni che possano giustificare comportamenti e in qualche modo avallare e dare una sponda. Oggi sappiamo quanto il linguaggio dei politici possa influenzare anche il clima

si parla di donne, infatti, all'interno dei *social* parte il rancore più esasperato ed è ancora più grave quando ci sono casi di femminicidio. Lo voglio dire in questa sede, soprattutto per le donne che fanno politica: capisco che la difficoltà

e quindi esprimo la solidarietà del nostro Gruppo a tutte le donne, a prescindere dalla collocazione politica. Questo è un punto importante, su cui noi maschietti dovremmo tutti "darci una regolata". Arrivo alla conclusione, parlando del coordinamento fra processo penale, civile e tribunale per i minorenni. Qui si può fare ancora un passo in avanti: ho parlato prima della corsia

sul versante penale non venga disallineata rispetto a una causa di separazione o di affidamento dei figli. Chiedo dunque, da questo punto di vista, un'attenzione e un equilibrio quando si legifera sull'affidamento dei figli e ogni riferimento il disegno di legge di Pillon non è puramente casuale.

che questa è una battaglia culturale prima ancora che politica e con la speranza che l'intensità del nostro impegno sia all'altezza della sfida, sia quando facciamo le dichiarazioni pubbliche che nella sfera privata, e con la consapevolezza che l'arma più importante che possiamo mettere in campo non passa da qui, ma passa dal racconto che facciamo ai nostri figli, dalle relazioni con le donne della nostra vita, dalla gentilezza dei nostri pensieri, delle nostre parole e dei nostri comportamenti.

non è la prima volta che in quest'Aula viene presentato un provvedimento contro la violenza sulle donne, non è la prima volta che viene affrontato questo tema. Se oggi ci troviamo nuovamente a votare una mozione su questa, che è una vera e propria piaga, significa che il problema continua purtroppo ad essere diffuso e di estrema attualità. Nei primi nove mesi del 2018, infatti, il numero delle donne uccise ammonta già purtroppo a 94 casi, ben 32 dei quali sono stati riconosciuti dalla polizia come casi di femminicidio. La violenza sulle donne non è un fenomeno che colpisce solo la donna in quanto tale, assumendo pertanto il carattere di violenza basata sul genere, ma mina l'uguaglianza e si pone come ostacolo allo sviluppo di una società democratica. La violenza nei confronti delle donne è una violazione dei diritti umani fondamentali riconosciuti e garantiti sia dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, sia dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Nonostante i numerosi strumenti di tutela e i progressi normativi attuati, anche a livello internazionale, per condannare e contrastare il fenomeno, continuano a purtroppo a perpetrarsi crimini contro le donne la cui trasversalità socio-economica e geografica ha indotto il Consiglio d'Europa ad adottare, nello specifico, la Convenzione sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica. La nostra mozione ricorda che nel 2013 il Parlamento italiano ha ratificato la suddetta Convenzione con la legge n. 77 dello stesso anno e ha approvato le disposizioni urgenti per il contrasto alla violenza di genere previste dal cosiddetto decreto antifemminicidio Quest'ultimo ha introdotto l'aggravante della violenza assistita, problema gravissimo appunto, per maltrattamenti commessi davanti ai figli ossia in presenza o in danno di un minore di anni diciotto, oppure in danno di persona in stato di gravidanza. quindi gli interventi legislativi repressivi e preventivi, tale fenomeno subisce continue recrudescenze. È indubbio che la violenza contro le donne abbia origini culturali e scaturisca principalmente dal fatto che l'uomo consideri la donna un suo possesso o un oggetto. pertanto necessario un intervento organico sui nostri giovani, che vanno educati fin dalla più tenera età: la scuola, in questo senso, ha un ruolo fondamentale: senza volersi sostituire alla famiglia, essa è chiamata ad avviare studentesse e studenti ad una riflessione sulla qualità dei rapporti tra uomo e donna, perché la nascita di una dialettica tra identità e diversità consente la più compiuta affermazione dell'individuo. Le istituzioni scolastiche devono dunque adottare opportune strategie di formazione, in collaborazione con le famiglie, le amministrazioni locali, i servizi socio-sanitari e tutti i soggetti dediti all'educazione e alla formazione. ricordiamo anche la relazione finale della Commissione parlamentare d'inchiesta sul femminicidio nella quale viene affermato che il problema è di entità tale da richiedere interventi che in termini di costi e rispetto dei vincoli di bilancio pubblico sono meno onerosi delle conseguenze derivanti dagli atti di violenza. Si tratta di interventi che includono anche il recupero degli uomini maltrattanti sotto il profilo del loro trattamento e della valutazione del rischio di recidiva. recidiva. Con la nostra mozione, impegniamo pertanto il Governo a fare quanto segue: adottare i provvedimenti necessari a promuovere e sostenere percorsi formativi all'educazione e al rispetto della donna; confermare, tra le politiche prioritarie dell'azione di Governo, il contrasto alla violenza; proseguire nella promozione di campagne d'informazione; intensificare iniziative e azioni di supporto, nonché percorsi di rieducazione degli uomini maltrattanti; adottare misure volte a rendere stabile e trasparente la destinazione delle risorse al finanziamento dei servizi e dei centri antiviolenza; infine, adottare ogni provvedimento necessario affinché le autorità giudiziarie possano accedere autonomamente per verificare l'eventuale iscrizione di procedimenti penali e civili per reati di violenza di genere. Signor Presidente, colleghi, non si può pensare di aver già fatto abbastanza. Il nostro pensiero e la nostra azione devono farsi sentire in maniera forte ogni giorno. Le donne oltraggiate necessitano di sentirsi sostenute e non lasciate sole; hanno bisogno di tanto coraggio, ma anche di tanta vicinanza. Facciamo sentire tutti insieme che ci siamo.

Presidente, colleghi, domenica scorsa ricorreva la Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza sulle donne, istituita nel 1999 dall'Assemblea generale dell'ONU. Venne scelto il 25 novembre perché in tale data, nell'anno 1960, tre delle quattro sorelle dominicane Mirabal vennero trucidate, perché colpevoli di essersi ribellate alla dittatura di Trujillo. Il loro nome in codice era *mariposas* (farfalle) e vennero uccise a bastonate. Da allora in Italia e nel mondo si è fatto molto per superare la cultura del maschilismo imperante che pervade la nostra società. Menzionerò qui la Convenzione per l'eliminazione di ogni forma di discriminazione della donna adottata nel 1979 dell'Assemblea ONU, entrata in vigore nel 1981 e ratificata in Italia nel 1985, che ha tra l'altro istituito un comitato con il compito di verificare lo stato di applicazione delle norme a tutela dei diritti delle donne. Cito inoltre la Convenzione di Istanbul del 2011, che per la prima volta ha creato un quadro normativo completo a tutela delle donne, giuridicamente vincolante a livello internazionale. Questa Convenzione, che è stata ratificata nella scorsa legislatura (nel 2013), ha introdotto modifiche al codice penale e al codice di procedura penale, inasprendo le pene - tra le altre cose Nonostante ciò, nonostante la predisposizione del Piano d'azione contro la violenza sessuale di genere, prevista dalla Convenzione da ultimo citata, e nonostante il Piano d'azione straordinario adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 luglio 2015, i dati sui reati contro le donne nel nostro Paese sono terrificanti. Negli ultimi dieci anni sono stati compiuti 1.750 femminicidi, più di 150 all'anno, quasi uno ogni due giorni; e la stragrande maggioranza di questi è avvenuta in contesti familiari. Nel solo 2017 ci sono state più di 2.000 sentenze definitive per violenza sessuale e più di 1.800 per *stalking*. Innumerevoli poi sono le denunce per maltrattamenti e lesioni; e questa è solo la punta dell'*iceberg*, dal momento che la statistica attesta che in nove casi su dieci la vittima non sporge denuncia. È evidente che questi dati sono il frutto di una cultura che non ha ancora fatto pienamente i conti con la tendenza di noi uomini a prevaricare sulle donne. La violenza è solo l'espressione più grave e più evidente del fenomeno: fanno parte di questo stesso problema anche gli insulti sessisti o o la tendenza ad affidare alle donne incarichi lavorativi di minor rilievo e meno remunerati. Eppure, le donne sono il pilastro della nostra società, non fosse altro perché sono tuttora prevalentemente dedite all'educazione e alla crescita dei nostri figli; dobbiamo averne cura. Il nostro Paese è certamente tenuto ad adottare tutte le misure utili a prevenire ogni atto di violenza nei confronti dei diritti dei diritti delle donne e a garantire una parità di genere effettiva - vorrei dire assoluta - che si estrinsechi in una totale uguaglianza di diritti, in una pari opportunità di scelta del tipo di vita che una donna decide di vivere, nella più totale autonomia e indipendenza, nonostante i figli. Non è giusto che una donna sia continuamente combattuta e ricattata tra la ricerca del proprio posto nella società e il fare la madre. La scelta di fare solo la madre o di non fare solo quello deve essere una scelta libera; ogni disparità di trattamento economico deve essere contrastata e combattuta, perché inficia l'indipendenza della donna e la espone così al rischio di comportamenti prevaricatori. Per fare ciò, è necessario innanzitutto cambiare la nostra mentalità, tuttora decisamente maschilista. Per capire a che punto la nostra società sia poco preparata a respingere episodi di prevaricazione di genere, basti ricordare che persino in questa Aula, nella scorsa legislatura, alcuni senatori si sono rivolti a colleghe con volgari gesti sessisti o con epiteti come *vaiassa*, che in napoletano significa serva, sguattera. In questa legislatura ho ascoltato con le mie orecchie un collega gridare in Aula a una nostra senatrice: «Torna in cucina». Purtroppo questi insulti sono trasversali, nessun Gruppo è esente, coinvolgono tutti: è proprio una questione culturale. È chiaro che un tale clima è indice di un problema non risolto, come del resto attesta l'ultimo rapporto consegnato al Governo a luglio 2017 dal Comitato costituito dalla Convenzione ONU del 1979 citata in precedenza, che ha indicato alcune delle lacune del nostro sistema. Tale rapporto ha indicato con chiarezza che occorre, innanzitutto, rafforzare la consapevolezza delle donne circa i loro diritti e i rimedi a disposizione per denunciare le violazioni. Da tale rapporto, inoltre, emerge la mancanza di coordinamento tra le componenti regionali e locali e di una chiara definizione dei mandati e delle responsabilità. Ancora, e soprattutto, occorre agire in maniera incisiva sulla scuola, per eliminare le discriminazioni attraverso l'educazione alla parità di genere sin dalla prima infanzia. Questo Governo, fin da quando si è insediato, ha cominciato ad agire per superare siffatti problemi. Vorrei ricordare che ieri il Consiglio dei ministri, con l'idea di rafforzare la legge n. 119 del 2013, ha approvato il cosiddetto codice rosso contro la violenza sulle donne. una norma che servirà ad abbreviare i tempi di reazione alle denunce delle donne per maltrattamenti, violenza sessuale, atti persecutori e lesioni connessi a contesti familiari o di convivenza. Sarà rafforzato il canale preferenziale già previsto dalla citata legge n. 119: la denuncia dovrà essere portata subito a conoscenza del pubblico ministero, che avrà tempi strettissimi (solo tre giorni) per sentire la denunciante. Inoltre, la polizia giudiziaria dovrà dare priorità alle relative indagini. Tuttavia, il MoVimento 5 Stelle, che - lo ricordiamo con orgoglio - ha la più alta percentuale di membri donne rispetto a qualunque forza politica di sempre chiede che sia fatto ancora di più su questo fronte. Ecco perché, con la nostra mozione, chiediamo che il Governo assicuri che i finanziamenti stanziati attualmente siano erogati regolarmente, senza ritardi, e siano vincolati all'assunzione di impegni precisi, attribuendo priorità e valutando i risultati. Chiediamo, inoltre, che vengano previsti indicatori per la valutazione dell'impatto degli stanziamenti. Chiediamo che venga predisposta una sezione, all'interno del sito del Dipartimento per le pari opportunità, per rendere accessibile la rendicontazione delle attività finanziate: neanche un euro deve essere sprecato. Chiediamo poi che si aggiorni la mappatura dei centri antiviolenza, anche per stimare il fabbisogno e adeguarne lo stanziamento. E ancora: chiediamo di assumere iniziative nell'ambito della scuola, educando alla parità e definendo linee guida che forniscano indicazioni per includere nei programmi scolastici i temi dell'educazione alla legalità e del contrasto alla violenza sulle donne. Chiediamo, ancora, che venga intrapreso un percorso che porti a iniziative di formazione degli operatori della giustizia, delle Forze dell'ordine e dei servizi sociali per affrontare il fenomeno; che si prevedano percorsi specifici in carcere per gli autori di violenza sessuale e di sfruttamento della prostituzione, compresa la destinazione di parte del reddito in favore del risarcimento della vittima, e si garantisca che le vittime di reati quali lo sfruttamento della prostituzione possano essere inserite in percorsi, al fine di rompere definitivamente il legame con gli sfruttatori. Chiediamo, quindi, ai colleghi di approvare tale mozione e al Governo di impegnarsi su tali obiettivi, affinché tutte le *mariposas* italiane, tutte le farfalle che si ribellano alle ingiustizie, non debbano più subire violenze o discriminazioni.

come ha già annunciato il collega che mi ha preceduto, l'Assemblea dell'ONU scelse la tragica, ma luminosa vicenda delle sorelle Mirabal per sollevarsi dal particolare all'universale, dal singolo caso di una violenza commessa barbaramente, alla violenza con la V maiuscola, che troppo a lungo ha dominato e domina i rapporti di genere, in virtù dell'impegno civile che esse dimostrarono. Ma non ci furono solamente impegno e coraggio nella loro tragica fine, bensì fragilità, impotenza e il sinistro marchio di un destino avverso. Nel suo romanzo «Un uomo», dedicato al compagno eroe della Resistenza al regime dei colonnelli greci, Oriana Fallaci sostenne di vedere in Alekos tutte le vittime da lei conosciute delle torture e dei soprusi dei totalitarismi, una dopo l'altra. Allo stesso modo noi oggi dobbiamo andare all'universale e vedere, ricordando le tre sorelle Mirabal, non solamente le donne vittime della violenza politica - e qui potremmo citare a proposito la nostra Norma Cossetto - ma tutte le donne di ogni età ed estrazione sociale che hanno subìto una qualsiasi forma di violenza. Purtroppo non è sempre possibile condannare con fermezza i soprusi subiti dalle donne, perché nel mondo contemporaneo, contraddistinto dai flussi di informazione globale, dalle tendenze e dai grandi portatori di interesse negli ambiti della comunicazione, certe forme di violenza sulle donne sono messe in secondo piano rispetto ad altre. La mozione n. 55 intende ristabilire una equità che ad oggi è mancata e accendere i riflettori anche su quelle forme di violenza che ideologicamente vengono tollerate, sottaciute e addirittura giustificate. In molti Paesi è tuttora tollerata la pratica delle spose bambine: giovanissime donne, minori di sedici anni, che vengono costrette a sposare un uomo molto più anziano di loro. È una forma di violenza aberrante, che definisce i rapporti di genere in forma preottocentesca e contribuisce a segnare uno scarto sostanziale tra i diritti civili goduti in Occidente e quelli goduti nei Paesi terzi. *(Applausi frequentemente accade che nei Paesi occidentali, compresa l'Italia, famiglie extracomunitarie lì residenti tornino al loro Paese d'origine per compiere, lontano dalla giustizia e dall'opinione pubblica dello Stato che li ospita, questo atto criminale. dai Gruppi L-SP-PSd'Az e M5S).* Un'altra pratica atroce, diffusa in molte parti del mondo, è la mutilazione genitale femminile, che costringe bambine e donne a essere cucite e poi scucite all'occorrenza, come bambole di pezza, in nome di un tradizionalismo miope totalmente incompatibile con i traguardi raggiunti dalla nostra civiltà. dobbiamo sottovalutare l'ipotesi che fenomeni simili si verifichino sottotraccia nelle città, nei quartieri e nelle campagne italiane. L'inclusione e la vigilanza attiva esercitata dai sistemi socio-sanitario e scolastico si confermano fondamentali a questo riguardo, perché anche questa è violenza sulle donne. Nell'Occidente postindustriale e interconnesso la pedopornografia è un fenomeno largamente diffuso, oltre che tristemente in diffusione, che mina drasticamente il corpo e l'anima di molte bambine sottratte alla loro innocenza e al loro diritto alla serenità individuale. La tolleranza deve essere zero verso chi usufruisce di materiale pedopornografico. *(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az)*. Oggi siamo in dovere di pretendere e patrocinare a gran voce la lotta contro costoro, perché anche questa è violenza sulle donne. Non dimentichiamoci inoltre che in alcuni Paesi occidentali, così come nella gran parte dei Paesi poveri, le donne, ricattate a causa della miseria e della fatica, sono costrette a vendere il loro stesso utero, offrendosi a sostenere la gravidanza di un figlio che non vedranno mai, che sarà strappato dalle loro braccia in nome dell'egoismo altrui e che, come in un supermercato, viene scelto, acquistato e ritirato. La parità di genere non sarà mai garantita finché l'utero in affitto rimarrà una pratica diffusa nel mondo e accettata da parte dell'opinione pubblica occidentale, perché anche questa è violenza sulle donne e direi anche sui bambini, perché non può essere precluso a un bambino il diritto ad avere la propria madre. Ancora oggi in Italia ci sono culture che considerano la donna antropologicamente inferiore rispetto all'uomo. Una figlia, una sorella e una moglie non possono scegliere come vestirsi, come autorealizzarsi, di chi innamorarsi, chi sposare, quanti figli avere, né esercitare attività per noi quotidiane come guidare l'automobile o intrattenere minime relazioni sociali. Anche in Italia - ripeto - è accaduto; probabilmente accade e tristemente continuerà ad accadere, nonostante tutti gli sforzi profusi dalle istituzioni. Quante ragazze che volevano vivere all'occidentale abbiamo pianto durante gli anni passati? Oggi parliamo anche dei loro ingiusti destini, perché anche questa è violenza sulle donne. L-SP-PSd'Az)*. Presidente, nel presentare questa mozione, vogliamo abbattere le barriere della discriminazione. Non vogliamo una serie A e una serie B delle donne vittime di violenza. Tutte hanno lo stesso diritto al ricordo. I loro destini bussano alle nostre porte per chiederci di fare qualcosa e la voce che possiedono è la stessa per ciascuna di esse, senza distinzioni. L'azione deve essere istituzionale, culturale, politica e anche avere di mira un unico grande nemico: l'ignoranza e l'intolleranza. La contrapposizione tra maschio e femmina è fuorviante e deleteria; non è l'uomo in quanto maschio a essere un pericolo per la sicurezza e la libertà delle donne, ma le idee e le istanze culturali nelle quali gli esseri umani tutti sono immersi.

Signor Presidente, penso che ciò di cui ci stiamo occupando oggi non sia un tema qualsiasi. E lo dico pensando al fatto che forse, anche oggi, avremmo dovuto utilizzare qualche grado in più di solennità, anche in questa Aula, e di maggiore attenzione rispetto a un tema che non riguarda soltanto la drammatica contabilità che ci troviamo a registrare ogni anno. Sono centinaia le donne uccise in quanto donne. Questo è il senso della parola femminicidio.

che siamo entrati nella fase della storia del mondo in cui si intravedono drammaticamente degli elementi comuni tra Paesi, tra quelle che abbiamo definito fino all'altro ieri democrazie consolidate o democrazie in transizione. Non è questa naturalmente la sede per analizzare questi elementi. Ce ne sono tanti: il mito della disintermediazione, un'insofferenza per la libera informazione e anche il vento di antipolitica che sta attraversando i Paesi occidentali, compreso il nostro. C'è una regressione sul terreno dei diritti, ma c'è un elemento che sta drammaticamente accomunando questi Paesi in tutto il mondo ed è un tratto machista e misogino del discorso pubblico,

corso dei mesi passati, quali «Dobbiamo obbligare le donne a partorire». Questa è violenza ed è esattamente la violenza che noi dobbiamo condannare e stigmatizzare.

una prima dimensione tutta culturale, che fa parte di come abbiamo costruito il nostro modello di società. Mi riferisco

ci sono gli elementi per poterlo fare. Alcuni interventi che mi hanno preceduto hanno fatto riferimento a ciò che è contenuto nella Convenzione di Istanbul; al fatto - ad esempio - che, a proposito della dimensione educativa del problema, l'articolo 24 prevede l'inclusione nei programmi scolastici di ogni ordine e grado di materiali didattici sulla parità tra sessi, ruoli di genere non stereotipati e il reciproco rispetto.

per i centri antiviolenza e per le case rifugio. Quelle risorse non possono e non devono essere toccate e, anzi, bisogna fare lo sforzo massimo affinché si possa fare un investimento serio su strumenti che hanno funzionato, possono funzionare e che tirano fuori molte donne dalla condizione di solitudine nella quale sono

per individuare in modo preventivo i casi di pericolosità. Molto spesso, infatti, le donne sono vittime di violenza e finiscono per essere ammazzate nonostante i tanti allarmi che esse stesse hanno lanciato nel tempo. Ritengo quindi che questo meccanismo debba essere messo a punto e reso

investire su questo terreno, e farlo velocemente. Noi dobbiamo fare dei passi in avanti sostanziali e dobbiamo farli in modo trasversale. Questo non può essere un elemento di battaglia politica, pur nel rispetto delle sensibilità diverse che potranno emergere. In tal senso, io mi auguro anche che l'istituzione della Commissione d'inchiesta sul femminicidio possa lavorare esattamente con questo spirito. E dobbiamo farlo alzando lo sguardo sul sul mondo, perché il tema del femminicidio, il tema della violenza sulle donne, riguarda sì le cosiddette civiltà avanzate - lo dico con un qualche elemento di ironia - come la nostra, ma riguarda anche molte altre realtà in giro per il mondo. Lo *slogan*

scomparse, sono state ammazzate e, molto spesso, mutilate. Quella giovane donna denunciava tale drammatica vicenda attraverso le sue poesie. È come se il potere avesse mostrato tutta la sua fragilità e avesse avuto paura della poesia. Noi dovremmo prendere esempio da questo. Dovremmo lavorare su questo tema con tutta la profondità che possiamo metterci perché, se lo facciamo, renderemo più forte la politica, renderemo più credibili le istituzioni e sicuramente renderemo più civile il nostro Paese. *(Applausi

Signor Presidente, è da venti anni che mi occupo della tematica della violenza contro le donne e mi sembra che si sia sempre allo stesso punto; anzi, a volte mi sembra che la violenza contro le donne sia aumentata. Questo è sicuramente dovuto anche al fatto che le donne non si vergognano più e trovano il coraggio per denunciare. Positivo è anche che la questione abbia guadagnato l'attenzione del dibattito pubblico. Venti anni fa era una tematica per poche donne che si battevano per i diritti, mentre oggi è l'intero Senato che discute della problematica e la maggior parte dei colleghi maschi ha preso coscienza di questa piaga sociale. Insomma, la questione è all'ordine del giorno della politica. Negli ultimi anni ci sono state innumerevoli convenzioni internazionali, a partire da quella di Istanbul, che obbligano tutti gli Stati a introdurre una serie di reati che puniscono la violenza sulle donne. Poi, notizia di queste ore, c'è anche il provvedimento cosiddetto "Codice rosso" emanato dal Consiglio dei ministri, che prevede la massima priorità per le denunce di violenza e l'obbligo del pubblico ministero di sentire la denunciante entro tre giorni. giorni. Se si sa quante donne vengono mandate a casa quando vogliono denunciare il marito, si comprende l'importanza di un provvedimento del genere. Nonostante tutto, i dati non sono incoraggianti. ore una donna viene uccisa. Nei primi otto mesi dell'anno, le Forze di polizia hanno raccolto denunce per ben 10.000 casi di maltrattamenti in famiglia, 8.500 per *stalking*, 3.000 per violenza sessuale. Tutto questo dimostra che ci vuole un cambiamento delle società, una decisa condanna di ogni forma di violenza verbale e fisica. Su questo chi rappresenta le istituzioni deve sempre dare l'esempio e invece non sempre accade, anzi: certi *post* di autorevoli esponenti politici si configurano come dei veri e propri inviti alla discriminazione di genere. Ma la violenza maschile è da ricondurre anche alla struttura sociale del potere. Fino a quando il rapporto tra i generi sarà segnato dalla disuguaglianza e dalla dipendenza, la violenza contro le donne sarà sempre presente. Sappiamo bene che tutto questo non è modificabile da un giorno all'altro e che ci vuole una convinta e radicale azione della politica, che non deve limitarsi solo alle parole ma deve prevedere atti concreti. Pertanto, con la nostra mozione chiediamo al Governo di rafforzare le misure cautelari introdotte con la legge del 2006; di investire nella formazione dei soggetti che operano a stretto contatto con le vittime di violenza come le Forze dell'ordine; di mettere a disposizione abbastanza fondi per i centri antiviolenza; di incentivare l'occupazione femminile, considerato che la dipendenza economica della donna rappresenta terreno fertile per gli uomini violenti; introdurre misure per incentivare la partecipazione dell'uomo al lavoro di cura della famiglia, introducendo un congedo parentale usufruibile solo dal padre e retribuito con un'alta percentuale del reddito. E, infine, data l'importanza dei *media*, chiediamo di introdurre strumenti finalizzati a vigilare sugli operatori della comunicazione, al fine di garantire una rispettosa rappresentazione della figura femminile.

a pubblicare - ognuno di voi - parole di scusa e soprattutto di dissociazione da certi pensieri che sono ignobili, che mi vergogno solo a ripetere (si parla di soffocare, si parla di ginocchia sbucciate). Non vi invito a vedere il *blog* dei 5 Stelle per rendervi conto della gravità

Signor Presidente, onorevoli colleghi, le mozioni all'esame dell'Aula sono l'ennesimo segnale che il Parlamento vorrebbe dare per affrontare e cercare di arginare l'ormai annoso problema della violenza sulle donne. Siamo in attesa dell'insediamento della Commissione di inchiesta sul femminicidio e a tal fine mi auguro che tutti i Gruppi diano quanto prima i nominativi delle senatrici e dei senatori che ne faranno parte,

in occasione della Giornata internazionale sulla violenza sulle donne. Ricordo con commozione anche il film «Red Land», che parla delle violenze ripetute, subite da una studentessa italiana, Norma Cossetto, violentata da 17 partigiani di Tito,

per affrontare e difendersi da ogni tipo violenza e per venire a conoscenza e usufruire dei servizi di aiuto presenti sul territorio nazionale. Sempre più donne in Italia decidono di dire basta e mettere fine alle violenze subite denunciando. Da gennaio a giugno di quest'anno il numero gratuito di pubblica utilità (1522), promosso dal Dipartimento per le pari opportunità diversi anni fa e gestito da Telefono Rosa, ha ricevuto solo a Roma 444 chiamate da parte di donne vittime di violenza, riuscendo in sei mesi quasi a raggiungere il numero totale di telefonate del 2017. L'aumento, d'altronde, è evidente anche nel resto d'Italia, dove sono arrivate quasi 5.000 telefonate. C'è quindi di sicuro un significativo aumento delle donne che chiedono aiuto e decidono di mettersi nella condizione di sperare di ricevere assistenza. però non vuol dire che siano aumentate le violenze: potrebbe voler dire che finalmente sta aumentando la capacità delle donne di reagire. Ed è un segnale molto positivo nella nostra battaglia contro il fenomeno sommerso della violenza, che dimostra una sempre maggiore consapevolezza delle donne che escono allo scoperto e trovano il coraggio di denunciare le violenze subite, che molto spesso avvengono all'interno delle mura domestiche. Sta poi a noi, però, dare una risposta in termini di sicurezza e protezione al loro coraggio. Il numero 1522 per chiedere assistenza e denunciare è sicuramente uno strumento importante, ma c'è ancora moltissimo da fare. Mi auguro a tal fine che il provvedimento approvato ieri in Consiglio dei ministri, il cosiddetto possa davvero portare lo snellimento delle procedure burocratiche delle denunce, che già si è sveltito, ma non abbastanza; di un *iter* giudiziario che da sempre chiediamo più breve. Mi auguro che finalmente le autorità giudiziarie possano accedere autonomamente in rete per verificare l'eventuale iscrizione di procedimenti penali per reati in tema di violenza e procedimenti civili per separazione e divorzio, nell'ambito dei quali sia necessario assumere determinazioni

l'assenza di conoscenza del tribunale dei minori che dà l'affido condiviso nei casi di maltrattamento in famiglia. I tribunali e le procure devono parlarsi e deve essere messa fine a questa situazione che lede i diritti alla sicurezza delle donne e dei loro figli. Per le vittime sono veramente tempi lunghi e massacranti: una tortura che deve aspettare a volte anni per arrivare a un provvedimento definitivo. Sarebbe ora anche di eliminare il rito abbreviato per il reato di femminicidio. Il cosiddetto "Codice rosso" dovrebbe inserire anche il patrocinio gratuito quando le associazioni di volontariato si costituiscono parte civile. sicuramente molto importante lavorare nelle scuole per un cambio di passo nella mentalità e per riabituare i nostri figli, fin da bambini, al rispetto della persona. Ho avuto il piacere di incontrare

di sensibilizzazione sul tema della violenza. Il ruolo della scuola e dell'università è fondamentale e queste sono le prime istituzioni che devono fare della prevenzione un principio cardine contro ogni violenza, anche perché purtroppo le statistiche ci dicono che l'età delle vittime è sempre più bassa e stiamo riscontrando anche una diminuzione dell'età degli autori di violenza. Infine, mi auguro che il Governo possa reperire già nella legge di bilancio per il 2019 maggiori fondi per i centri antiviolenza, a favore di tutte quelle vittime che hanno avuto il coraggio di denunciare e hanno certamente necessità di ricostruire la propria vita.

la sua battaglia per l'adozione di bambini da parte di coppie omosessuali per occuparsi di un problema impellente e urgente come quello del femminicidio e della violenza sulle donne. *(Applausi

*(PD)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la violenza sulle donne rappresenta una tra le più gravi violazioni dei diritti umani e la più diffusa tra quelle perpetrate nel nostro Paese. di una dimensione di cui assumiamo progressiva consapevolezza a partire proprio dalla stratificazione dolorosa ed eterogenea di vissuti che si manifestano ormai quasi quotidianamente in tutta la loro efferatezza. La storia ci mette di fronte a queste situazioni, evidenziando anche il rischio di un'assuefazione o addirittura di una resa da parte della collettività. Ora il tema è esploso fino a spingere la legge a contrastare il fenomeno e a responsabilizzare lo Stato a prendere una posizione netta. Nell'educazione, nella formazione, nel lavoro e nelle relazioni sociali e professionali le donne continuano a essere in molti casi, anche silenziosamente, sottilmente penalizzate attraverso il rovesciamento simbolico di pseudoforme di gratificazione che, piuttosto, privano le stesse dei territori della libertà vera e dell'autodeterminazione. Si evitano il clamore, la discriminazione rumorosa e i divieti altisonanti, tutto questo perché non è ancora stata cancellata la secolare convinzione che alla donna spetti un posto altro, un ruolo altro, una funzione altra. Questo atteggiamento si perpetua nei linguaggi, nei metalinguaggi, negli usi del fare sociale e, soprattutto, attraverso una comunicazione e un'informazione, anche commerciale che, come abbiamo evidenziato nella nostra mozione, è deleteria della dignità della persona, stigma di un abbassamento del livello culturale e valoriale. La discriminazione ha attraversato indenne decenni di appannata sensibilizzazione, scarsa educazione, a tratti anche inefficace legislazione. Oggi noi, eletti dal popolo, non possiamo nasconderla e soprattutto non possiamo nasconderci di fronte a essa. Abbiamo il dovere morale, civile e storico di imprimere una svolta definitiva; abbiamo l'obbligo di intervenire con vigore e fermezza, con un'azione che significhi tutta la volontà e la forza dello Stato, soprattutto - consentitemi di dirlo - squarciando il velo di Maya dell'ipocrisia che circola nelle ripetute e certe volte pericolosissime pronunce di buone intenzioni, tante volte destinate a restare tali (cioè solo pronunce), in questo modo sollevandoci dalla responsabilità di tenere il punto fermo sulle condotte e sulle scelte politiche da mettere in campo. dare alle donne e agli uomini un segnale deciso e univoco, che parta da questo Parlamento e arrivi a rassicurare ciascuna di noi e tutti del fatto che lo Stato è con noi. A tal fine, occorre affrontare politicamente il tema partendo dalle cause che lo generano, che sono di carattere culturale. Tra di esse vi è il tema della solitudine e della sofferenza irrisolta, perché laddove la sofferenza è irrisolta e inascoltata essa diviene la giustificazione di una spinta che deborda nel terreno della violenza. L'antecedente del femminicidio è il conflitto che affonda le sue radici nella condizione di irrisolutezza che la solitudine e l'incomunicabilità generano. Sono questioni sociali che necessitano di azione politica. Pensiamo alle soluzioni, ma pensiamo anche ad attivare sentinelle sociali, intervenendo sull'educazione e sulla sensibilizzazione - soprattutto delle giovani generazioni, ma non solo - per lo sviluppo di una consapevolezza piena del dramma che si ripete. Lo Stato deve dare sostegno e supporto a tutte le donne che sperimentano le conseguenze infami dell'ignoranza e dell'indifferenza e deve farlo ben prima che queste sfocino nella violenza domestica e nel femminicidio. È fondamentale riflettere e agire sulle strutture "Codice rosso" illustrato ieri rafforza la nostra convinzione che servono misure di stampo securitario, ma il vero tema oggi è quella dell'attuazione delle leggi e, soprattutto, soprattutto, delle risorse finanziarie messe a disposizione. Un atteggiamento opaco da parte di chiunque può rappresentare drammaticamente una palude livida, una zona d'ombra, che a noi oggi tocca svelare e attraversare, dando forma e voce reale a scelte politiche sostenute da passione e da piena responsabilità. Oltre ogni giornata, nel dispiegarsi del *krónos* e del *kairós*, il tempo per noi tutti deve essere quello pieno del rispetto.

molte persone ritengono che questi momenti di riflessione siano inutili, che siano solo parole. Secondo me non è affatto così: sono momenti per ragionare e per ribadire che ci sono

È normale usare certe espressioni e considerare bonariamente un commento sessista o un complimento troppo pesante.

che è venuta meno in questi anni. È successo che i genitori non sono più autorevoli e i figli si permettono di mancare loro di rispetto;

Non possiamo pretendere di fare una legge e di tornare improvvisamente autorevoli: dobbiamo riprenderci l'autorevolezza come politici, come parlamentari, come genitori, come mogli, come mariti, come insegnanti e così via. È comporta un costo personale, però è solo grazie a questo processo che possiamo pensare di trasmettere ai giovani un messaggio giusto.

fragilità emotiva e il non controllo degli impulsi. Tutti noi proviamo rabbia, gelosia e tutte le emozioni possibili e immaginabili,

cittadini stranieri, che mi è stata detta in Libia nel 2005 da una bravissima guida, che mi ha detto: «Vedi, c'è un problema, perché tutto ciò

anche attraverso l'approvazione del provvedimento cosiddetto "Codice rosso", che costituisce un grandissimo passo avanti, per il quale ringrazio immensamente il Governo, il ministro Salvini e anche il nostro ministro Bongiorno, che da anni si batte su questi temi.

Riteniamo che, in un contesto come quello di oggi e, soprattutto, su un argomento così importante come quello di oggi, non sia corretta la strumentalizzazione per attacchi politici. Il MoVimento 5 Stelle ha sempre condannato fermamente qualsiasi tipo di atteggiamento sessista e maschilista a danno delle donne e quindi non accettiamo critiche da forze politiche che forse non sempre hanno dimostrato rispetto delle donne. Tuttavia ci fa piacere che alcune donne si siano rese conto di questa cosa. Procedo con il mio intervento. In occasione della giornata contro la violenza sulle donne, che ricorre il 25 novembre, l'ISTAT ha svolto per la prima volta un'indagine sui servizi offerti dai centri antiviolenza in Italia. I dati diffusi dall'Istat sono a dir poco allarmanti. Nel 2017, quasi 50.000 donne si sono rivolte almeno in un'occasione ad un centro antiviolenza per denunciare molestie, maltrattamenti, insulti, aggressioni o peggio. Entrando nel dettaglio dei numeri forniti dall'istituto statistico, emerge ad esempio che su un totale di 49.152 donne, che nel 2017 si sono rivolte ai centri finanziati dalle Regioni, il 59,47 per cento ha iniziato un percorso di uscita dalla violenza,

dati inquietanti, tanto più se incrociati con quelli diffusi dall'Eures, secondo il quale nei primi dieci mesi del 2018 in Italia ci sono stati 106 femminicidi, uno ogni tre giorni. I centri forniscono in prevalenza servizi di ascolto e accoglienza, supporto legale, orientamento e accompagnamento ad altri servizi, supporto psicologico, aiuto nel corso di allontanamento dal *partner* violento, orientamento lavorativo e sostegno all'autonomia: in alcuni casi, il servizio è fornito direttamente dal centro; in altri, in collaborazione con i servizi sul territorio; in altri ancora, il centro assolve la funzione di indirizzamento. Continuando a leggere i dati forniti dalla relazione dell'ISTAT, si scopre che la maggiore parte dei centri (quindi l'85,8 per cento) lavora in rete con altri enti del territorio e che quasi tutti (il 95,3 per cento) aderiscono al numero verde nazionale 1522 contro la violenza e lo *stalking*. *stalking*. Sono circa 4.400 le operatici che nel 2017 hanno lavorato presso i centri antiviolenza, il 56,1 per cento delle quali è stato impegnato esclusivamente in forma volontaria. Le figure professionali presenti nei centri sono operatrici specificamente formate. Il 93 dei centri antiviolenza prevede una formazione obbligatoria e nell'85 per cento dei casi è il centro stesso ad aver organizzato i corsi di formazione per il personale. I centri antiviolenza sono nati in Italia grazie al lavoro del movimento delle donne e all'esperienza dei consultori che, a supporto della legge sull'interruzione volontaria di gravidanza, hanno permesso diffusamente alle donne d'incontrarsi tra loro, per prendere per prendere parola su corpo, sessualità, relazioni con gli uomini e quindi, di conseguenza, sulla violenza e sugli stupri subiti in famiglia, oltre che nei contesti amicali e lavorativi. Ai centri antiviolenza si rivolgono donne di tutte le provenienze sociali e la classe più rappresentata è quella media. Riguardo alla violenza sulle donne, spesso si dimentica che sono gli uomini ad esserne protagonisti: la violenza è un problema maschile e, a parte alcuni casi sporadici, gli uomini non si sentono direttamente chiamati in causa a discuterne. I centri antiviolenza rappresentano quindi un laboratorio privilegiato per osservare e registrare i cambiamenti nelle relazioni di genere: attuano campagne di educazione al rispetto e alla differenza nelle scuole e con gli adolescenti, secondo la logica di prevenire nei giovanissimi la diffusione di comportamenti violenti e stereotipati.

sulle nuove generazioni si debba lavorare, quindi che, ancora una volta, la grande responsabilità ricada sui concetti di educazione e rispetto, partendo dalle basi, dalle nuove generazioni e dalla prevenzione. Questa frase mi piace dirla con senso di amore: insegniamo ai bambini la delicatezza dei gesti il garbo dell'anima; insegniamo alle bambine a volersi bene; insegniamo il rispetto con il rispetto, l'amore con l'amore e la non violenza con la non violenza, perché i bambini seguono ciò che facciamo, più di ciò che diciamo. *(Applausi

come molti hanno già ricordato, secondo le stime più prudenti, milioni di donne hanno subìto almeno un episodio di violenza nel corso della loro vita e, solo in Italia, almeno un milione e mezzo è stata vittima di stupro. Anche se negli ultimi anni le cose fortunatamente stanno migliorando, ancora troppe poche donne denunciano, soprattutto nel caso di violenza domestica. Non lo fanno per paura, per vergogna e probabilmente anche perché non godono di quella autonomia economica

Casi di cui si parla troppo poco, in ossequio a un malinteso politicamente corretto e in ossequio a un relativismo culturale che noi denunciamo e condanniamo nel modo più assoluto. Troppe donne, dicevo, non denunciano perché vengono lasciate sole dopo la denuncia; troppe donne vengono uccise dal loro aguzzino perché lasciate sole dallo Stato. È facile, cari colleghi, dire alle donne di denunciare, senza chiedersi perché così poche ancora lo fanno, senza chiedersi perché ancora, parte delle Forze dell'ordine, ci sia una sottovalutazione della violenza contro le donne, soprattutto se questa avviene all'interno delle mura domestiche, e senza chiedersi come mai, anche nel caso in cui la magistratura emetta dei provvedimenti di protezione, questi troppe volte restano grida manzoniane, provvedimenti senza concreta efficacia e senza concreta attuazione.

che ha escluso l'aggravante dello stupro di gruppo nei confronti dei carnefici di Desirée, soltanto perché - pensate un po' - i suoi carnefici, dopo averla resa incapace di comprendere cosa succedeva e di difendersi, la stupravano a turno anziché tutti insieme. Ecco, sono decisioni come queste, cari colleghi, che allontanano le donne dalla volontà di denunciare. *(Applausi dai pur nel rispetto della separazione dei poteri, di stigmatizzare queste decisioni, che così gravemente influiscono sullo stato d'animo delle donne che vogliono affrancarsi dalla loro condizione di soggezione, da loro condizione di sudditanza e dalle violenze che troppo spesso devono subire, non soltanto violenze fisiche, ma anche psicologiche, economiche e sul posto

quel manifestante che ha sputato addosso a un poliziotto nell'esercizio del suo dovere. Sono decisioni che allontanano l'opinione pubblica e i cittadini dal senso delle istituzioni. Abbiamo sentito ieri l'annuncio del Governo e speriamo che per una volta non ci si fermi soltanto agli annunci. Siamo d'accordo, finalmente, sull'adozione di una corsia preferenziale per certi reati, dai maltrattamenti in famiglia allo *stalking*, alla violenza sessuale. Siamo soprattutto d'accordo sull'obbligo del pubblico ministero di sentire la vittima di questi reati entro settantadue ore, in modo che le Forze dell'ordine che ricevono le denunce non le mettano in un cassetto, non se ne dimentichino e non le sottovalutino. Ecco perché, cari colleghi, Fratelli d'Italia sostiene con convinzione la mozione che ha presentato come prima firmataria la collega Isabella Rauti.

sono di gran lunga di più i punti di contatto che le differenze presenti tra le mozioni. Se già partissimo da questo nodo cruciale, che è un nodo di condivisione profonda, per proporre al Governo, attraverso la sua proposta del codice rosso, la possibilità di creare un ponte tra un'iniziativa di tipo governativo e una di tipo parlamentare, condivisa,

scritte e presentate da donne, anche se fortunatamente sottoscritte da molti colleghi dei rispettivi Gruppi; sono la rappresentazione di un sentire comune e condiviso. È questo sentire ciò che deve costituire il vero punto di cambiamento di un sistema. Dico questo per una ragione molto semplice. Noi abbiamo delle leggi. La legislatura precedente, di cui sono felice di aver fatto parte, è intervenuta più volte. Abbiamo cominciato, all'inizio della legislatura, con una famosa mozione sul femminicidio;

siamo andati avanti, in diversi altri passaggi, sempre con questo sentire comune di denuncia. Non sto qui a ricordare ai colleghi quante volte, negli interventi di fine seduta, si è sollevato il caso, il problema, la concretezza del singolare rispetto a una sofferenza più ampia e più generale. Tuttavia, questo non alimenta affatto la speranza, l'ottimismo, una prospettiva di fiducia in un futuro che si sia tradotto, nei fatti, in una riduzione degli episodi di violenza. A volte mi chiedo se la violenza che con maggiore frequenza occupa le prime pagine dei giornali e i telegiornali a ripetizione, per diverse serate di seguito, non sia il frutto di una maggiore conoscenza, che rende più esplicita la denuncia, o non vi sia l'emulazione, che nasce

fa il rettore dell'università di Harvard sosteneva che il cervello femminile fosse inferiore come capacità. Detto dal tempio della cultura, dove sono nati tantissimi premi Nobel, questa aggressione al femminile risultava francamente svalutante. Ma ancora di più mi ha sorpreso, pochi mesi fa, dall'università di Pisa, che rappresenta uno dei templi della cultura, una delle eccellenze tra le università italiane, l'affermazione dell'inidoneità della donna ad affrontare gli studi scientifici, cosa assolutamente falsa; viceversa, i fatti dimostrano quanto la donna sia impegnata in tutti i lavori e in tutti gli studi di stampo scientifico. Questo, sempre che si voglia tenere conto del contributo positivo che la donna dà e non si voglia denunciare, invece, quella forma di violenza, il famoso

la presenza reale di ciò che c'è, ma anche il contributo specifico, in termini di qualità relazionale, di rapporto, di capacità di costruire reti di comunicazione. Infine, una piccola notizia comparsa l'altro giorno sulla prima pagina del «Corriere della sera»: sembra che a Milano ci siano decine e decine di monumenti a uomini illustri e non ce ne sia neppure uno a una donna. Questo avviene a Milano, noi siamo a Roma, non vogliamo metterci in discussione, ma intanto è una cosa che colpisce.

passare sotto silenzio quella che invece è la violenza che si scatena nell'arroganza, nella presunzione, nella convinzione di poter imporre un lessico, una scala di valori, un criterio di giudizio che tenga sostanzialmente la donna in una posizione subordinata, senza mai riconoscere al femminile la sua specificità, il suo valore, la sua forza, la sua capacità di trasformare il contesto. *(Applausi

ogni aggiornamento dei dati statistici, che sono impressionanti e che sono già stati citati negli interventi che mi hanno preceduto, ci confermano che questo orrore di aggressività fisica, psicologica e sessuale è in aumento e che i maltrattamenti domestici, anche contro le donne in gravidanza, anche di fronte ai figli terrorizzati, sono sempre più diffusi. La maggior parte di questi femminicidi sono commessi da uomini che avevano un rapporto sentimentale con le loro vittime. Un rapporto sentimentale: ma di quali sentimenti stiamo parlando? Questo è uno dei nodi più importanti, forse quello da cui partire, come è stato già accennato. Mi riferisco all'analfabetismo emotivo, alla mancanza di parole, all'incapacità di dare nome a ciò che proviamo e quindi di attuare dei comportamenti conseguenti a ciò che si prova. Certamente la prima emergenza, citata in tutti gli interventi, è quella di combattere i costi umani, sociali ed anche economici della violenza sulle donne; far applicare le leggi, potenziare i centri antiviolenza, accompagnare le vittime verso percorsi di autostima e coraggio. l'azione più importante è la prevenzione. Partiamo allora dal potenziare un grande investimento educativo, già iniziato nella scorsa legislatura, che coinvolga la scuola e non solo, fin dalla prima infanzia, sull'uso delle parole, dei libri di testo, dei giochi, dello sport, della scelta degli studi, dell'impegno sociale, per far crescere bambini e bambine nel rispetto delle differenze di genere e della pari dignità. Perché crescere negli stereotipi sessisti discredita la stima delle donne in quanto persone, penetra nelle relazioni familiari, nei rapporti di lavoro, nei percorsi di carriera. Due, allora, sono in particolare gli obiettivi che vorrei sottolineare: l'educazione socio-affettiva e l'educazione alla corporeità. Assumete la responsabilità di voi stesse. Questo la scuola, dove non lo fa la famiglia, dovrebbe insegnare alle ragazze per favorire lo sviluppo di un autentico progetto di sé, in un sistema patriarcale che le svaluta, le umilia, le ferisce, dove la violenza verbale e lo *hate speech* in rete aprono la strada anche alla violenza sul corpo. È arduo contrastare l'immaginario, l'immaginario, che è come uno specchio deformante alimentato dai *media,* che spinge ad esibire un corpo, ridotto a oggetto, strumento di desiderio, possesso di qualcun altro. Il rischio è che le ragazze vengano allora espropriate di un vissuto del proprio essere un corpo. Dunque, assumere la responsabilità del proprio corpo-persona significa insegnare alle ragazze che possono essere forti come Bebe Vio e perfino esplorare lo spazio, come Samantha Cristoforetti. Educare alla dignità del corpo femminile fa, quindi, parte dell'educazione alla differenza nel cammino di crescita verso l'autenticità, ma per arrivare a questo occorre che gli educatori (uomini e donne) siano convinti del valore femminile. Si tratta di un compito non facile che che coinvolge parallelamente anche lo stereotipo maschile. I bambini possono imparare da educatori autorevoli che si può essere ugualmente virili senza uniformarsi al modello tradizionale della forza fisica, della durezza e della competitività. È, dunque, tempo di insegnare ai ragazzi che, per esempio, la tenerezza può essere oggi una nuova virtù eroica. eroica. Presidente, la conclusione politico-pedagogica è, quindi, un apparente paradosso: essere uguali per poter essere diversi perché il valore dell'uguaglianza resta irrinunciabile, ma ogni differenza è una risorsa e senza pari dignità questa differenza rimane opposizione, inferiorità e dipendenza. Bisogna, quindi, educare avviare nuovi comportamenti, valori e modalità di comunicazione, dove l'incontro con l'alterità di genere si ponga come luogo del noi, dove ci sia un rapporto autentico da un tu a un altro tu in una differenza dove la contrapposizione, che caratterizza i rapporti tradizionali, possa tradursi in uno scambio che cresce nella reciprocità di parole e di comportamenti.

prima di tutto vorrei rivolgere un ringraziamento ai senatori del mio Gruppo che unitamente hanno firmato questa mozione che pone l'attenzione su tutte le forme di violenza che ogni giorno le donne subiscono in Italia e nel mondo. I dati della violenza sulle donne parlano chiaro: più di 700 milioni di donne si sono sposate quando ancora non avevano compiuto diciotto anni e di queste circa 250 milioni hanno preso marito addirittura prima dei quindici Sono 120 milioni le bambine che hanno subìto violenza sessuale; per non parlare del fenomeno delle mutilazioni genitali, a cui sono costrette ancora 200 milioni di donne in ben 30 Paesi, dove questa pratica è considerata una tradizione da rispettare. In Italia ogni settantadue ore muore una donna vittima di femminicidio e una donna su tre ha subìto almeno una volta violenza. Qualcuno potrebbe stupirsi di questi dati, perché spesso il termine violenza viene associato esclusivamente alla sua forma più estrema, il femminicidio. Invece, le forme di violenza nei confronti delle donne sono molteplici: donne umiliate, maltrattate, lese nell'autostima o, ancora, ostacolate nel raggiungimento dell'indipendenza economica; donne alle quali viene vietato di decidere liberamente e autonomamente della propria vita, donne alle quali viene offerto del denaro per partorire e donare ad altri un proprio figlio. In quest'Aula qualcuno pensa ancora che sia giusto farlo. Il parto è l'atto d'amore più grande; è il miracolo che un uomo e una donna creano. Non può essere altro, non quello che una certa parte politica vuole farci credere essere uguale perché vendere il proprio corpo è solo violenza. Una donna che, infatti, dà il proprio utero lo fa per soldi, nient'altro. Le conseguenze psicologiche che ne conseguono non vengono spesso prese in considerazione. Se i numeri non mentono - non mentono e ne siamo certi - tra queste donne ci sono nostre vicine di casa, amiche e conoscenti e ci potrebbero essere anche le nostre bambine. Gli Stati hanno il dovere di esercitare la responsabilità dovuta per prevenire, indagare e perseguire gli atti di violenza contro le donne. Gli Stati hanno il dovere di perseguire e punire i responsabili degli abusi e delle violenze e, a differenza del Governo precedente che non ha presentato alcun disegno di legge *ad hoc* ma solo linee guida, questo Governo proprio ieri ha dimostrato, ancora una volta, che è passato dalle parole ai fatti. Proprio ieri, il Consiglio dei ministri, infatti, ha firmato il disegno di legge "Codice rosso" a tutela della donna e contro la violenza sulle donne, nato dall'iniziativa della Fondazione Doppia Difesa. Troppe donne, infatti, nonostante le denunce, muoiono o continuano a subire maltrattamenti in attesa di giudizio. Con questo disegno di legge, invece, chiediamo un intervento immediato e diretto. Entro tre giorni le donne dovranno essere ascoltate, la polizia giudiziaria dovrà comunicare immediatamente al pubblico ministero le notizie di reato acquisite, senza lasciare discrezionalità sulla sussistenza dell'urgenza. Tra i vari punti previsti, infatti, c'è la modifica dell'articolo 347 del codice di procedura penale che stabilisce l'obbligo della Polizia giudiziaria di comunicare immediatamente al pubblico ministero le notizie di reato acquisite, se riguardano delitti di maltrattamenti, violenza sessuale, atti persecutori e lesioni aggravate, commessi in contesti familiari o di semplice convivenza, senza lasciare discrezionalità sulla sussistenza dell'urgenza. Vi è poi la modifica dell'articolo 362, che prevede che nei casi di violenza domestica e di genere il pubblico ministero proceda all'ascolto della vittima del reato entro tre giorni dall'avvio del procedimento. C'è l'integrazione dell'articolo 370 che obbliga la Polizia giudiziaria a dare priorità allo svolgimento delle indagini delegate dal pubblico ministero, quando si tratta di reati di maltrattamenti e violenza sessuale, atti persecutori e lesioni aggravate, commessi in ambito familiare o di semplice convivenza. Al contempo le risultanze acquisite con l'attività svolta devono essere documentate e trasmesse in modo altrettanto tempestivo al pubblico ministero, Il disegno di legge introduce infine l'obbligo di formazione per la Polizia di Stato, Arma dei carabinieri e Polizia penitenziaria, attraverso la frequenza di corsi presso specifici istituti, da fornire al personale coinvolto in procedimenti in materia di violenza domestica e di genere. Le donne tutte devono essere poste nelle condizioni di cogliere il pericolo, denunciarlo e rivolgersi alle istituzioni competenti e da queste ricevere efficace e tempestiva tutela. quindi un appello alle donne: denunciate, non abbiate paura, lo Stato finalmente c'è ed è al vostro fianco con ogni mezzo a sua disposizione. che, al contrario di quanto è stato dichiarato da chi mi ha preceduto, noi non facciamo alcun taglio. Lo ha dichiarato proprio ieri il presidente del Consiglio Conte; non solo nuove regole, ma anche finanziamenti e sono già stati recuperati, dal precedente stanziamento, 33 milioni di euro per il 2019 per un fondo di emergenza *ad hoc*, coordinato dal sottosegretario alle pari opportunità Vincenzo Spadafora. importante quindi che il decreto-legge arrivi finalmente e velocemente in Senato e alla Camera, dove mi auguro (ma sono certa sarà così) verrà votato all'unanimità perché, come detto inizialmente, non può esserci colore politico in queste lotte. Pertanto il mio augurio è che le donne possano ricevere maggiore tutela a nome di tutti noi. *(Applausi dai

la nostra mozione ha al suo interno alcune iniziative molto semplici, ma concrete, volte a trasformare in fatti le tante parole che abbiamo ascoltato in questi giorni. Giorni in cui si è discusso di femminicidio, in cui il Paese si è fermato a riflettere; giorni ai quali dobbiamo far seguire azioni, perché abbiamo il dovere di fornire strumenti di contrasto e prevenzione che non restino esclusivamente *slogan*. La violenza di genere purtroppo non è un fenomeno eccezionale e non può essere affrontato una sola volta all'anno. Ieri è stato approvato dal Consiglio dei ministri il codice rosso per velocizzare l'*iter* delle denunce delle donne vittime di violenza. Un utile strumento di contrasto che deve essere affiancato però ad altre misure, come anche sostenuto dagli organismi internazionali. Il rapporto delle associazioni di donne sull'attuazione della convenzione di Istanbul in Italia, che analizza la situazione italiana in materia di contrasto alla violenza sulle donne, ha evidenziato che nel nostro Paese la normativa esistente in concreto non viene applicata e che ancora, malgrado le risorse economiche stanziate e le azioni messe in campo per affrontare il fenomeno, la distribuzione e l'applicazione disomogenea delle stesse risorse sul territorio nazionale fa sì che la tutela dei diritti delle vittime di violenza non sia effettiva. Con questa mozione oggi vogliamo rendere possibile che quanto stanziato annualmente per i centri antiviolenza e le strutture di accoglienza per mamme e minori sia erogato regolarmente, senza ritardi e vincolato all'assunzione di impegni precisi, all'individuazione delle priorità e alla valutazione dei risultati ottenuti. È necessario colmare le lacune di applicazione delle leggi in materia, introducendo modalità di attuazione volte a snellire i procedimenti con chiara individuazione della norma ed imposizione della stessa. Dobbiamo confrontarci con le associazioni che lavorano da anni su questa difficile tematica e con i centri antiviolenza nelle loro varie declinazioni per comprendere meglio non solo le questioni strettamente legate agli episodi che si verificano quotidianamente, ma l'impatto degli stanziamenti economici e puntualizzare strategie di intervento efficaci. La mappatura dei centri antiviolenza, anche con il necessario supporto del Dipartimento per le pari opportunità, deve essere aggiornata a cura del Governo secondo i *report* ricevuti da Regioni e Province autonome, in modo da stimare il fabbisogno reale di questi centri e garantirne, non solo la sopravvivenza, ma soprattutto un funzionamento appropriato, in grado di assicurare servizi adeguati su tutto il territorio nazionale. È fondamentale poi agire in campo educativo, perché il problema è prioritariamente culturale, garantendo il diritto delle bambine, soprattutto e in particolar modo, di studiare per avere una parità di opportunità e di diritti e contribuire così all'inclusione sociale ed economica delle future donne. Quindi, intervenire predisponendo percorsi di formazione per chi opera nei settori educativi; potenziare i progetti scolastici mirati a offrire pari opportunità di relazione e di inserimento nella vita sociale ed economica delle donne; attuare campagne informative all'interno delle scuole, ma anche in ogni ambito lavorativo, volte a diffondere la cultura della non violenza e del rispetto del prossimo; attivare formazione specifica e, in alcuni casi, anche obbligatoria in ogni settore professionale coinvolto nelle attività di prevenzione e di contrasto alla violenza di genere; assumere iniziative di comunicazione intelligente che non si limiti solo per fare maggiore presa sull'opinione pubblica a enfatizzare la donna vittima, fuorviando la percezione dell'immagine femminile, ma faccia emergere il meraviglioso mondo femminile. Quindi, insisto in quest'Aula, senza ritenerlo scontato, su un impegno fattivo del Governo ad assumere ogni decisione contro qualsiasi atto di violenza contro le donne. Infine, concludo, rivolgendomi, da donna, parte di una metà del cielo, a quell'altra metà del cielo, che mi piace pensare siano gli uomini, i nostri figli, i nostri mariti, fidanzati, amici, colleghi, padri, invitandoli a indignarsi per ogni episodio di violenza contro le donne, a testimoniare i modelli di relazione positiva tra uomo e donna, ad uscire dal silenzio dimostrando, finalmente, il rispetto per le loro figlie, le loro mogli, le loro fidanzate, le loro amiche, le loro colleghe e le loro madri. Trovino in se stessi, e noi mamme in questo abbiamo grande responsabilità, la forza culturale ed etica di rapportarsi alle donne sempre in termini di uguaglianza solidarietà

Sono dei giovanissimi, ai quali credo sia rivolta una sia rivolta una considerevole parte dei nostri interventi. Interventi che mi permetto di chiosare dicendo che tocca soprattutto a noi uomini, a noi padri,

la discussione. Comunico che sono state presentate le riformulazioni delle seguenti mozioni:

Signor Presidente, restituiamo a questa discussione la solennità che merita, soprattutto per la presenza di giovanissimi che, effettivamente, saranno coloro che porteranno avanti i valori che costruiamo insieme qui oggi.

A nome del Governo intervengo per dire che la lotta alla violenza sulla donne è la partita di tutti. Questo è il *claim*, per nulla retorico, dello *spot* realizzato dalla RAI per il Dipartimento delle pari opportunità in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne del 25 novembre. Spero sia davvero la partita di tutti, a prescindere dagli schieramenti politici. Vorrei rassicurare sulla questione fondi: il Governo non ha diminuito i fondi destinati alle iniziative per contrastare la violenza sulle donne. A parte un taglio MEF ordinario e ricorrente del 2,7 quest'anno saranno messi a disposizione 33 milioni di euro che saranno tutti finalizzati ad azioni concrete per prevenire e proteggere le donne e punire veramente i colpevoli. Finché resterà in carica questo Governo, fondi dello Stato saranno investiti nei centri antiviolenza e nelle case rifugio, come da riparto stabilito assieme alle Regioni, e anche in iniziative concrete e di sicuro impatto per le vite di migliaia di donne vittime di violenza nel nostro Paese. Due fondi in particolare sono allo studio: in primo luogo un fondo *ad hoc*, equo e duraturo, in favore delle vittime affinché ricevano, immediatamente dopo la violenza subita, un effettivo sostegno economico.

dove ospitare le donne vittime di violenza nella fase intermedia, che va dalla denuncia alla presa in carico da parte dei centri antiviolenza. Il 26 settembre scorso il sottosegretario Spadafora ha istituito e convocato la prima riunione della nuova cabina di regia politico-programmatica prevista dal piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2017-2020 al fine di dare concreta attuazione al piano Il piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne, adottato dal Governo precedente, riprende i contenuti della Convenzione di Istanbul, ma necessita di concretezza e operatività per evitare la frammentarietà e la sovrapposizione degli interventi. Solo la stesura di un piano operativo in cui sono declinati gli obiettivi in azioni e interventi specifici con l'indicazione di tempi, modalità e risorse, è in grado di dare concretezza alla strategia. Proprio in questa direzione la risposta del Governo tutto, e in particolare dei diversi ministeri competenti oltre alle Regioni e agli enti locali, è stata positiva e si è concretizzata. Il 21 novembre scorso c'è stata, appunto, la seconda riunione della cabina di regia politico-programmatica con l'adozione di un primo piano operativo. La collaborazione con le principali associazioni e con le parti sociali si è concretizzata grazie alla loro partecipazione al comitato tecnico istituito il 25 ottobre 2018 che costituisce il braccio operativo del piano strategico nazionale contro la violenza degli uomini il Consiglio dei ministri ha approvato un disegno di legge, il cosiddetto "Codice rosso", che ha come obiettivo quello di garantire una corsia preferenziale, ovvero una maggiore tutela alle vittime di maltrattamento e violenza sessuale, atti persecutori e lesioni commessi in contesti familiari o nell'ambito di relazioni di convivenza, assicurando la tempestività dell'adozione degli interventi cautelari o di prevenzione. Credo di aver delineato un impegno convinto e concreto che il Governo porterà avanti con estrema determinazione. Mi auguro che questo avvenga con il contributo di tutti.

Il Gruppo per le Autonomie voterà a favore di tutte le mozioni, con la sola eccezione di quella a prima firma Pucciarelli. Non si può classificare la violenza di genere come un fatto che riguarda il terzo mondo o «alcune culture presenti anche nel nostro Paese», come è scritto nella mozione. Inoltre, se si vuole qualificare la maternità surrogata come forma di violenza contro le donne, si deve parlare molto prima dello sfruttamento della prostituzione, che invece non viene menzionato;

E non sfugge neanche la tipica frase antifemminista secondo cui bisogna uscire da dinamiche di contrapposizione tra i sessi, come se la violenza fosse figlia di un conflitto tra uomo e donna e non una forma di prevaricazione di un sesso sull'altro. Infine, in quella mozione non si dà alcuna rilevanza al tema della parità di genere come requisito per prevenire l'insorgere della violenza. Si sa che la maggior parte dei femminicidi avviene nella fase della separazione. Pertanto, ci vuole un diritto di famiglia che rafforzi la posizione della donna e che non la indebolisca, come invece purtroppo accade con la proposta Pillon. Per quel che riguarda le altre mozioni, ho sentito tante prese di posizione appassionate e competenti, anche da parte di colleghi maschi, che ringrazio personalmente. Così come sono state espresse tante buone idee, che spero davvero trovino centralità nell'azione del Governo e del Parlamento. Le migliaia di donne che hanno manifestato sabato scorso a Roma, insieme alle tante manifestazioni che si sono svolte in tutte le città italiane, ci dicono che su questo tema sta maturando una importante consapevolezza, a cominciare proprio dalle donne. Anche in Parlamento ci sono state tutta una serie di iniziative di sensibilizzazione che vanno nella giusta direzione. Adesso non bisogna mollare la presa, ma far sì che questa maggiore consapevolezza si trasformi in atti concreti, in misure per promuovere la parità di genere e per debellare quest'orrenda piaga sociale.

le mozioni che stiamo per votare affrontano un tema drammatico, che non può certo essere al centro della nostra attenzione solo in occasione di celebrazioni e ricorrenze. Io ho sempre sostenuto che quella contro il femminicidio e la violenza di genere non possa e non debba essere una battaglia solo delle donne, ma un impegno di tutti coloro - uomini e donne - che credono nell'uguaglianza, nella tutela dei diritti della persona, nella democrazia. Ogni condotta che mira ad annientare la donna nella sua identità e libertà, non solo fisicamente ma anche nella sua dimensione psicologica, sociale e lavorativa, è una violenza di genere. È un fenomeno che ha tante forme: dal sessismo di certe affermazioni considerate a torto leggere, alle offese, alle minacce; dall'uso, che purtroppo sta diventando frequente anche nel nostro Paese, dell'acido come forma di sfregio, fino ai troppi casi di femminicidio. Ci sono donne che subiscono quotidianamente maltrattamenti, violenze sessuali e psicologiche, minacce e molestie e non dobbiamo dimenticare che molte delle vittime di omicidio o di lesioni gravi avevano già denunciato episodi di violenza e di maltrattamento. Altre, invece, non avevano mai chiesto aiuto per sfiducia nelle istituzioni, per mancanza di mezzi o per una pericolosa sottovalutazione delle violenze subite. Donne che, trovata finalmente la forza di uscire da situazioni di questo tipo, non incontrano poi il sostegno sociale e istituzionale necessario per ricostruire la propria vita. «Non è normale che sia normale» è uno *slogan* che rende meglio di ogni altra cosa questa situazione. Per contrastare efficacemente questa deriva ritengo essenziale garantire alle vittime una protezione efficace sin dai primi atti penalmente rilevanti.

Forse si dovrebbe anche incrementare la formazione delle Forze di polizia o istituire sezioni specializzate e sezioni anche nelle procure della Repubblica, come già alcuni uffici di procura fanno. fanno. Bisogna consentire di prevenire le offese ulteriori più gravi che, con un crescendo di intensità, spesso culminano nell'omicidio; inoltre, si dovrebbe facilitare l'emersione di sopraffazioni, che in troppi casi vengono tenute nascoste dalle stesse vittime per paura o vergogna. Prendiamo atto che il Governo ha presentato con grande enfasi il cosiddetto disegno di legge "Codice rosso" per le donne vittime di maltrattamenti. Voglio ricordare che un intervento in tal senso esiste già ed è stato approvato nella scorsa legislatura con la legge 15 ottobre 2013, modo, ricordo che esiste già l'obbligo per le Forze di polizia che ricevono una denuncia di trasmetterla immediatamente alle procure. Occorre l'impegno a mettere in pratica tutto ciò e non certo i soliti *slogan*. Iniziate a lavorare per far funzionare le cose. La ratifica della Convenzione di Istanbul segna un progressivo aumento di interventi e norme di grande importanza, trattandosi del primo strumento giuridicamente vincolante che predispone un quadro giuridico completo di protezione contro le violenze. L'innovazione più rilevante consiste nell'individuare nella prevenzione e protezione delle vittime il perno delle strategie di contrasto, anche attraverso azioni preventive nel settore educativo e dell'informazione, nonché misure di sostegno medico e psicologico. Questo obiettivo richiede l'impegno di tutte le forze del Paese per educare e informare i cittadini, a partire dalle scuole, sottraendo le vittime al bisogno economico e sostenendo il miglioramento delle condizioni di vita delle donne e l'uguaglianza giuridica e di fatto. È necessaria una reazione di condanna forte e chiara. Non esistono tolleranza, né giustificazione alcuna per le condotte che ledono i diritti delle donne. La consapevolezza condivisa della gravità

Stiamo finalmente mettendo in discussione i nostri antichi modelli di riferimento e, in questo senso, la scuola ha un ruolo decisivo nell'insegnare fin dalla più tenera età che non esiste scusante, non ci sono eccezioni, alibi o giustificazioni a comportamenti che violano la libertà di una donna. Stiamo cercando, finalmente, di far abbandonare la cultura che prevedeva ruoli fissi e immutabili, ma nel profondo - sappiamolo - ci sono ancora stereotipi e gabbie che vanno sradicate. La cronaca è veramente colma di storie dove uomini di tutte le età usano la violenza, nelle sue diverse forme, contro le donne. Quello che desta ancora più allarme è che per ogni storia di cui abbiamo notizia ce ne sono altre, molte altre, in cui il dolore e la violenza vengono a volte dal silenzio, dalla vergogna e, purtroppo, dall'impunità. Fondamentale in questo senso è il sostegno da parte dello Stato, in tutte le sue articolazioni, ai centri antiviolenza, ai centri di ascolto e di accoglienza su tutto il territorio nazionale. Della mi avvio a concludere - non devono dunque parlare anche gli uomini, ma soprattutto gli uomini. Troppo a lungo si è sbagliato approccio: per anni abbiamo lasciato le donne sole a combattere questa battaglia di civiltà. Oltre ai numeri ci sono le persone: anche un solo episodio è di troppo. Quindi dobbiamo continuare senza sosta a parlarne, per cambiare i comportamenti sbagliati sin da subito.

A chi rappresenta i cittadini viene chiesto di essere conseguente nei voti, nelle azioni, nelle decisioni, nei provvedimenti. Essere contro la violenza di genere significa non esporre donne, nello specifico addirittura minorenni, alla gogna dei *social,* come ha recentemente fatto anche il Ministro dell'interno. Centinaia di commenti indegni si sono riversati su tre giovanissime studentesse senza che il titolare del profilo ne prendesse le distanze. Essere contro la violenza di genere significa aumentare le tutele economiche, lavorative, sociali e familiari nei confronti delle donne, nel contesto familiare e anche nei casi di separazione e di divorzio. Per questo nessun voto e nessuna mozione serviranno, se contestualmente non verrà ritirato il disegno di legge Pillon, bocciato senza alcuna riserva anche dal sottosegretario con delega alle pari opportunità Vincenzo Spadafora, del vostro stesso Governo. È con queste motivazioni che annuncio il voto favorevole del Gruppo Misto-Liberi e Uguali alla mozione a prima firma della senatrice De Petris.

Detto questo, però, colgo l'occasione, perché mi piacerebbe fare un appello a tutte le donne dell'Aula, a tutte le colleghe. Credo che per quanto riguarda la violenza

poche volte durante l'anno, ma sicuramente in concomitanza del 25 novembre, della Giornata mondiale contro la violenza sulle donne - non rendiamo un servizio per risolvere o almeno tentare di risolvere

Anzi, lasciatemelo dire, care colleghe, siamo un po' strumento, ci facciamo utilizzare per essere forma e molto poco sostanza. Fedeli)*. Cari colleghi, prendete allora il coraggio a due mani: portate all'interno del vostro mondo una riflessione. Vedete voi di diventare protagonisti su questo tema. Credo che noi donne abbiamo soltanto una possibilità di aiutare voi uomini, e dovremmo farlo meglio e forse di più, nel nostro ruolo di madri. di madri. Sono mamma di un figlio maschio e l'unica cosa che ho cercato di fare - poi è tutto da vedere se ci sarò riuscita - è quella di educare mio figlio all'amore. cosa che noi donne possiamo fare, in qualità di madri, è educare i figli maschi all'amore, ad amare le donne, le donne, perché l'amore porta con sé il rispetto, che molto spesso manca in voi uomini. Non sono parole mie, ma si è sempre detto che il grado di civiltà di una popolazione è misurato dal grado di rispetto che gli uomini hanno nei confronti delle donne. donne. Care colleghe, sottraiamoci dunque a questo teatrino che tutte le volte ci vede protagoniste. Oggi non sono contenta di essere qui a fare la dichiarazione di voto: lo dico onestamente. Forse avrebbe dovuto farla un uomo al posto mio e, allo stesso modo, stamattina avrei voluto sentire parlare molti uomini, che invece, tolte alcune eccezioni, non ho sentito. Colgo anche l'occasione per parlarvi di un'altra cosa: capisco che non siamo e non sono di moda, perché non sono e non siamo politicamente corretti,

2.783 atti di violenza contro le donne nella nostra nazione, 1.115 sono stati commessi da chi italiano non è.

Questo ci dovrebbe interrogare e far diventare un po' tutti politicamente scorretti, perché è vero che molte violenze sessuali si commettono all'interno delle nostre famiglie, è vero che ciò riguarda anche molti fidanzati e mariti italiani - è tutto molto vero

perché quegli uomini che hanno ammazzato e stuprato Desirée non avrebbero dovuto essere sul territorio nazionale. La seconda questione è molto legata alla sicurezza, perché ricordate che molto spesso più sicurezza vuol dire più libertà, soprattutto per noi donne. questa giornata a Desirée proprio perché volevamo far notare l'enorme problema che l'immigrazione incontrollata ha portato nella nostra nazione.

prendere coscienza, perché sin quando non prenderemo coscienza di questo tema non porteremo alcun contributo per risolvere un problema così grave e di cui si parla da così tanti anni.

753 stupri hanno visto coinvolte ragazzine che non avevano compiuto

di stuprare e violentare persone che non sono maggiorenni, che hanno quattordici anni. Lo stupro di gruppo è fatto all'interno di uno schema tribale ben definito.

a fronte di un magistrato che cerca di derubricare il reato di stupro, come nel caso di Desirée,

l'altro? Non possiamo dunque tapparci gli occhi né non voler vedere come l'immigrazione incontrollata - o meglio l'invasione, per chi è politicamente scorretto - abbia aumentato i casi di violenza sulle donne.

Fratelli d'Italia voterà a favore di tutte le mozioni, ma vogliamo sottolineare a tutti i colleghi di aprire gli occhi e non essere troppo politicamente corretti.

vari passaggi e sul tratto di fondo dell'intervento che mi ha preceduto. *(Applausi dal Gruppo PD).* Lo dico senza alcuna polemica, perché credo che oggi lo sforzo debba continuare ad essere quello di costruire un clima e una tensione unitari su un tema che abbiamo scelto di affrontare

per rinnovare con essa un impegno a continuare sul percorso per sconfiggere il drammatico fenomeno della violenza sulle donne. Molte cose sono state dette in quest'Aula oggi; voglio esprimere una parola sincera di apprezzamento per i tanti uomini che sono intervenuti, a partire dal mio collega Alfieri e dalle sue parole. E molte cose sono state dette in questi giorni alla Camera, nel dibattito che ci ha preceduto, e anche sulla stampa, nel dibattito pubblico. Sarebbe quindi forse davvero superfluo ripetere ancora numeri e statistiche drammatiche e tristi, che ovviamente non vanno mai dimenticate, perché sono un punto essenziale di riferimento e, per quanto drammatiche, hanno un loro portato e una loro forza. Sono numeri però che ci inchiodano tutti a una grande responsabilità: la lotta alla violenza sulle donne e a tutte le forme di violenza sulle donne è e deve continuare a essere una priorità per tutti, da giocare per forza di cose insieme. E allora oggi un impegno credo sia prioritario: niente retorica e niente polemica politica sulla pelle e sul corpo delle donne. Niente, dal Gruppo PD)*. La valutazione però deve essere lucida e attenta della portata enorme di un fenomeno che continua a emergere nella sua atroce drammaticità. Tutti i dati ci raccontano di un fenomeno ampio, diffuso e purtroppo strutturale. Ecco perché - e lo dico in premessa con molta chiarezza - non credo siano state utili e sagge le parole del sottosegretario Spadafora - che conosco anche come persona attenta a questi temi e che mi sarebbe piaciuto vedere qui in Aula stamattina - in occasione della celebrazione del 25 novembre. A lui al Governo diciamo che gli avversari non siamo noi, non sono le vostre opposizioni. Se questa è la vostra battaglia, noi siamo dalla stessa parte e chiediamo a voi di essere al nostro fianco. Dobbiamo intenderci, però, su quale sia il nostro comune avversario. Per noi è rappresentato - lo dico con chiarezza - da un'organizzazione patriarcale della società, ancora troppo spesso fondata su una profonda, iniqua e ingiusta disparità di poteri tra uomini e donne. È questa disparità che fa da incubatore a rapporti e relazioni squilibrate e malate, che generano sopraffazione e violenza. violenza. Voglio ricordare a me stessa e a tutti noi che la violenza è il primo strumento con cui si afferma il dominio fisico e culturale degli uomini sulle donne, quel dominio che in questo secolo è stato messo in discussione, per fortuna, da tante conquiste, da diritti inviolabili e sociali delle donne, che però in nessuna democrazia, una volta raggiunti, possono dirsi raggiunti per sempre. Per questo voglio tornare al nostro ruolo. La nostra qui in Parlamento non può che essere un'alleanza, il nostro deve essere uno sforzo unitario e coeso per stanare tutti i tentativi espliciti e reconditi di difendere o ricostruire modelli di società, per fortuna in gran parte superati, fondati su ruoli profondamente diversi e squilibrati tra uomini e donne. Sono questi gli avversari e i nemici di questa battaglia. Ecco perché il Partito Democratico ha lavorato e sperato di poter costruire una voce condivisa intorno a una mozione unitaria. Dobbiamo riconoscere che questo terreno non è ancora del tutto condiviso; c'è chi ha scelto di mantenere elementi divisivi. Noi però non ci arrendiamo. Noi voteremo a favore di tanti dispositivi e chiediamo di proseguire soprattutto sui punti di convergenza. In questi anni, e non solo negli ultimissimi, tanti risultati sono stati raggiunti, seppure in contesti politici e culturali molto diversi; anche in quelli che potevano apparire più ostici, si è sempre trovato lo spazio per fare passi significativi in avanti. Lo si è fatto da parte del Governo Berlusconi, con i provvedimenti sullo *stalking*, fino ad arrivare ai nostri ultimi Governi, che hanno impresso una decisa accelerazione a questo percorso. Potrei fare un elenco lunghissimo delle cose fatte: i piani antiviolenza, le case rifugio, i finanziamenti, la Convenzione di Istanbul, i protocolli delle Forze dell'ordine, il ministro Fedeli con il suo lavoro nel settore della formazione, le forze di polizia, anche dentro il percorso del processo. Voi ieri avete fatto un ulteriore passo e noi lo riconosciamo; non abbiamo problemi a riconoscere che anche piccoli passi, come quello compiuto ieri, vanno nella direzione giusta. Ovviamente valuteremo se ci saranno le risorse necessarie per rendere quegli impegni effettivi. Noi non vogliamo che ci venga riconosciuto il merito di tutto quanto fatto, non siamo qui per questo. Non ci vogliamo dividere su questo. Vi chiediamo però una cosa: proseguite sulla strada

Non possiamo perdere tempo, perché siamo preoccupati. Siamo preoccupati dal numero ancora troppo alto di comportamenti scorretti, atti persecutori, aggressioni e violenze mortali contro le donne. Molti comportamenti rimangono nascosti o non denunciati. Abbiamo denunciato un problema che riguarda innanzitutto la conoscenza delle situazioni in cui le violenze accadono, facciamo ancora troppa fatica a risalire alle dinamiche che ne sono all'origine. Per migliorare servono politiche di prevenzione larghe, che prevedano punti di riferimento a disposizione delle donne che avvertono questa difficoltà. Siamo preoccupati perché non vediamo portare avanti l'azione per attuare il piano nazionale approvato nel 2017. Siamo preoccupati perché vediamo fermi i protocolli sulla formazione, quelli già firmati la polizia penitenziaria e la polizia municipale. Siamo preoccupati perché non vediamo passi in avanti per quanto riguarda il dialogo con il Consiglio superiore della magistratura. Su questo punto il senatore Alfieri è già stato chiaro.

e sembrare inopportuna, ma sono già passati oltre tre minuti dal tempo che le era stato concesso. La prego di concludere. VALENTE *(PD)*. Di fronte a un Ministro che fomenta senza remore la gogna pubblica contro tre giovani che lo avevano contestato si doveva levare l'indignazione di chi ha responsabilità di Governo su questo fronte. In ogni caso, ci preoccupa di più una cultura che sta ispirando tanti dei vostri provvedimenti. Non mi riferisco soltanto a una tendenza repressiva e punitiva, ma anche a una cultura giustizialista e forcaiola, che in nome di un tribunale del popolo e della giustizia, finisce per piegare diritti individuali, garanzie, libertà, rischiando così di minare alla base i princìpi fondamentali di uno Stato di diritto. Il PD vuole tenere il tema della violenza sulle donne fuori dalla contesa e dalla legittima battaglia politica. Vogliamo costruire su questo un terreno di lavoro comune. Lo vogliamo fare a partire dalla prossima sessione di bilancio. La faccio concludere, ma deve concludere, senatrice. VALENTE *(PD)*. Ecco perché io ho timore davvero che, guardando solo al fenomeno finale, quello su cui si interviene con la repressione quando il danno già è fatto, si commetta un grave errore; non basta per risolvere un problema, che è sociale prima ancora che penale, e non basterà aumentare le pene o inventarsi un'applicazione per mettersi il cuore in pace. Un Paese più sicuro per donne e uomini sarà un Paese dove libertà, diritti, autonomia, capacità di autodeterminazione saranno tutelate come proprie scelte di vita da parte di uno Stato non oppressore ma regolatore e garante di questi spazi di libertà. Credo che diritti e libertà delle donne misurino il grado di civiltà e progresso di un Paese. Il nostro compito è allora quello di arrestare qualsiasi tentativo di tornare indietro. Noi siamo pronti a fare la nostra parte e chiediamo a tutti di farla insieme a noi.

lo fece in onore delle tre sorelle Mirabal. Da uomo, da italiano e da ciociaro, quando immagino di legare il dolore di una donna a una data, non posso non pensare al 1944, quando, a seguito dello sfondamento della linea Gustav, i soldati marocchini *goumier*, incorporati all'esercito francese, furono ignobilmente ripagati dal generale Juin con un macabro regalo: cinquanta ore di assoluta libertà *(Applausi un vero e proprio diritto di preda, ossia il diritto di poter abusare liberamente e a piacimento di tutte le donne, di tutte le età, come fossero giocattoli di sfogo (le marocchinate). Sono date lontane, ma le ferite devono rimanere sempre aperte e indelebili, per rispetto, per capire, per non giustificare e per non dimenticare. Ancora oggi serpeggia il maledetto concetto di sudditanza, di sottomissione da imporre alle donne; una sottomissione che nasce da una cultura ignorante, cattiva,

e M5S)*. Disprezzo per il valore della gravidanza, non più un giustificato atto voluto e desiderato coscientemente, anche a tutti i costi, ma calcolato e comprato, servendosi della povertà economica di chi vende o deve vendere il proprio utero; disprezzo che sfoga nella volgare, distorta, malata ed egoistica soddisfazione della pedopornografia *(Applausi egoistico e superbo, che sfocia in violenza fisica, che troppo spesso e troppo facilmente porta a ferite indelebili, come quella dell'acido, o ad una morte che poi lascia morire i cari e i familiari Disprezzo che vuole giustificare offese e violenze psicologiche e spesso il mezzo di tale disprezzo è il telefonino, che si trasforma in una pistola silente, i cui proiettili micidiali ed anche mortali sono le parole, le offese, le minacce. registrati 1.827 casi di *stalking* e questo dato (in difetto se si considerano le resistenze, la paura, la vergogna e la bugiarda speranza del «non sia vero») impegna il Governo all'attenzione, alla correzione, al controllo di un atteggiamento della cultura del «se non sei mia non sarai di alcun altro». Si tratta di un atteggiamento malato che nel 2017 ha causato almeno 2.018 sentenze definitive di violenza sessuale e ha ucciso una donna ogni due giorni. L'85 per cento delle vittime sono familiari ed amanti. Eh sì, la morte ha le chiavi di casa per molte, troppe donne. Dispiace constatare in questi ultimi anni e non voglio essere tacciato di razzismo o frainteso in questo senso - anche il disprezzo della donna bianca. Purtroppo è una verità che impegna il Governo a non voler più ospitare bestie che uccidono senza pietà e senza paura abituati a riti e culture di un mondo che non ci appartiene. «Ho una bianca da stuprare»; è questa la frase di chi ha picchiato, sprezzato, accoltellato il corpo di una ragazzina di appena sedici e che poi l'ha scuoiata, spezzata, giugulata con una tecnica tipica di tradizioni religiose o culturali arretrate, la macellazione. sarà quindi un Governo che non accetterà queste bestie e che non vorrà mai dare un premio, una giustificazione o una riduzione della pena. Insegniamo ed obblighiamo al rispetto delle donne. «Amate e rispettate la donna, non cercate, in essa, solamente un conforto ma una forza, un'ispirazione, un raddoppiamento delle vostre facoltà intellettuali e morali. Cancellate dalla vostra mente ogni idea di superiorità, non ne avete alcuna». Sono parole di Giuseppe Mazzini. La donna non è uno strumento di piacere, un gioco, un vizio, un peso. La donna è l'inizio dell'avvenire. La donna siete tutte voi, senatrici che onorate quest'Aula. La donna è Liliana Segre. La donna è Silvia, la nostra volontaria rapita in Kenya; le donne sono Michelle e Giulia della fondazione Doppia difesa; donne sono le nostre madri e le nostre figlie. Noi della Lega, con tutti voi, coscienti delle difficoltà, siamo obbligati a difendere fino alla morte il rispetto morale, culturale, psicologico e fisico di tutte le donne. Per questo chiedo sincera collaborazione per provvedere alle disposizioni della Convenzione di Istanbul: prevenire violenze, proteggere e sostenere le vittime, perseguire i trasgressori, contrastare le violenze. Non sottovaluteremo la volontà di innescare un vero e forte cambiamento, di educare cittadini, di proseguire con la promozione di adeguate campagne d'informazione, rieducare gli uomini maltrattanti, aggiornare le mappature dei centri antiviolenza e aiutare le donne a capire che la sola amica non basta a salvarle. Può essere uno sfogo momentaneo, ma ci si deve affidare alle Forze dell'ordine, che in questi ultimi anni stanno aprendo degli sportelli necessari e importanti per la difesa delle donne. Ieri, il 28 novembre, abbiamo dimostrato l'impegno al rispetto alle donne con l'approvazione da parte del Consiglio

Non facciamone perciò una gara; evitiamo, anche perché perdereste. Onoriamo l'impegno e lavoriamo piuttosto, come abbiamo fatto la scorsa settimana, quando il nostro Capogruppo della Lega ha organizzato un convegno

Governo, colleghi e colleghe, innanzitutto ringrazio i colleghi e le colleghe di ogni schieramento per la sensibilità dimostrata sul tema e in particolare - mi si consenta, senza battute - le colleghe del PD per l'immediata condivisione di un percorso che, pur nelle reciproche differenze di impostazione, ci ha visto collaborare fattivamente. Signor Presidente, Governo, cari colleghi e care colleghe, il rispetto della dignità umana e della persona costituisce il bene primario di ogni democrazia e di ogni azione politica.

La violenza sulle donne invece, anche nei Paesi più evoluti tra cui il nostro, ancora persiste, insiste e nonostante la messa in campo di ogni iniziativa legislativa possibile, aumenta. La violenza sulle donne è il fenomeno più democratico che esista e il più cosmopolita, quindi non si può circoscrivere. È un fenomeno subdolo, strisciante, di cui troppo spesso ci si rende conto solo quando portato alle estreme conseguenze. La violenza sulle donne ha mille facce *stalking*, *mobbing*, maltrattamenti, percosse, molestie, sfruttamento sessuale, riduzione in schiavitù, discriminazione, coercizione, menomazione, differenze salariali e violazione dei diritti, femminicidio. Ecco, il Femminicidio, questo neologismo che riesce sempre a far discutere. Consentitemi un inciso prima di entrare prima di entrare nel merito: personalmente sono contraria a ogni forma di «femminilizzazione» dei ruoli perché secondo me le funzioni non hanno genere. Il Presidente del Senato rimane il Presidente (uomo o donna che sia) come il Sindaco o il Ministro rimangono il Sindaco e il Ministro, uomini o donne che siano ma, invece, reagisco quando sento polemizzare su questo termine da parte di persone che non riescono a vederne la differenza rispetto all'omicidio. In questo caso la differenza c'è, eccome, nel momento in cui la violenza estrema contro una donna si compie da parte dell'uomo verso una donna in quanto donna, in quanto femmina, nella accezione più negativa e sbagliata di oggetto di possesso!

là dove comunque ci sia ancora la concezione della donna percepita sesso debole, nel senso che la debolezza fisica, la maggiore o la diversa sensibilità sono considerati i limiti che, in menti grette e ignoranti, rendono lecite azioni spregevoli nei loro confronti. E il «là dove» non è purtroppo solo dall'altra parte del mondo ma anche «qui e ora» nella nostra civilissima Europa, nella nostra civilissima Italia, da Nord a Sud senza differenze. Perché oggi siamo ancora qui a sollecitare il Governo con una mozione? Perché oggi siamo ancora qui a manifestare, a portare testimonianze, a manifestare, a portare testimonianze, a sensibilizzare in ogni modo? Siamo ancora qui perché nonostante tutti gli sforzi, tutte le leggi e tutte le manifestazioni i numeri diffusi dalle statistiche sono impressionanti: solo in Italia ogni due giorni e mezzo viene uccisa una donna. E i

l'OMS la considera la più vergognosa e la più pervasiva. Tanto da considerarla un flagello sociale, la prima causa di morte delle donne fra i sedici e i quarantaquattro anni. Ecco perché oggi siamo ancora qui a parlarne. Per arrivare a non doverne parlare più. In Italia, sono stati nel tempo introdotti numerosi strumenti di civiltà e tutela femminile, a partire dalla riforma del diritto di famiglia nel 1975 quando finalmente la donna

alla legge del 2009 contro lo *stalking* o a quella del 2006 che vieta le pratiche di mutilazione genitale femminile. Ci sono però reati che ancora vanno codificati nel nostro ordinamento: nuove fattispecie di reati subdoli, striscianti e pericolosissimi: per esempio pene severe per chiunque pubblica o divulga attraverso strumenti informatici, informatici, telematici o digitali immagini e video privati sessualmente espliciti senza il consenso delle persone rappresentate. Alle azioni dirette alla rivoluzione culturale devono poi aggiungersi ulteriori interventi sul piano legislativo, perché alla gravità di questo fenomeno si può davvero rispondere soltanto con provvedimenti articolati. Dobbiamo spingere per un sistema di prevenzione organizzata,

denunce, indagini più rapide sui casi di violenza alle donne e l'obbligo per i pm di ascoltare le vittime entro tre giorni e corsi di formazione per le forze di polizia. L'iniziativa è più che lodevole ed è la sintesi di quanto da sempre richiesto in maniera trasversale, ma ricordo che se a quanto enunciato non segue un impegno economico preciso ed immediato all'interno della legge di bilancio, l'enunciazione rischia di rimanere soltanto un proclama. proclama. La rivoluzione culturale deve tradursi in una presa di coscienza collettiva della società, che deve poi trasferirsi, come stiamo tentando di fare, in una battaglia comune di uomini e donne contro questa grave realtà. Le rivoluzioni costano; non sono costi, ma investimenti; e allora cambio termine: il Governo deve investire, investire e investire, perché l'investimento produrrà un rientro. Investire sulla scuola e sull'educazione, come migliore garanzia perché la scuola è un osservatorio privilegiato.

È ora di andare oltre. Come leggevo in uno dei tanti messaggi che in questi giorni sono girati sui *social*, e qui vi prego di prestare attenzione: «Viviamo in una società che insegna alle donne a difendersi dallo stupro invece di insegnare agli uomini a non stuprare le donne». E in questo, come hanno ricordato più colleghe, le madri dei figli maschi siamo noi donne ed è quindi nostro primo dovere. Ecco perché la richiesta della mozione rispetto alla necessità di un obbligo per gli uomini maltrattanti di seguire un percorso di riabilitazione presso centri specializzati. Un intervento a parte e specifico (lo faremo poi e spero che riprenderemo questo punto) meriterebbe poi l'orribile questione degli abusi sulle donne con disabilità. Sono il 36 per cento le donne disabili vittime di violenza, il doppio delle altre donne. È agghiacciante! E l'orrore aumenta se si pensa che, nella maggior parte dei casi, chi commette violenza su di loro è proprio chi dovrebbe prendersene cura. Mi viene la pelle d'oca. L'introduzione delle telecamere di sorveglianza negli istituti si rivelerà fondamentale e ringrazio per questo l'iniziativa della nostra collega Gabriella Giammanco.

In quest'Aula oggi con emozione e come sprone lasciatemi rileggere l'articolo 3 della nostra Costituzione: «tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

condivisa che ci deve vedere tutti alleati che deve essere vinta stando fianco a fianco anche in memoria di tutte le donne cadute sul campo. Signor Presidente, onorevoli colleghi, quante volte la giustificazione ad un atto di violenza commesso tra le mura domestiche, e più raramente fuori di esse, è: «Lo faccio perché ti amo troppo». Una frase che può apparire banale ma che, in realtà, il più delle volte nasconde dolorosi retroscena. Quelli che, in questi giorni in particolare, abbiamo sentito palesati nei racconti delle tante donne che, purtroppo, vanno ad arricchire le statistiche sulle molestie, sullo *stalking*, sulle violenze e - fatto più grave - sul femminicidio. Domenica scorsa si è celebrata in tutto il mondo, come già avete ricordato tutti, la giornata dedicata a questo terribile fenomeno. Ebbene, non basta alleggerirsi la coscienza con un solo momento celebrativo. Proprio perché insieme a storie terribili abbiamo ascoltato tante opinioni, a volte viziate dalla poca conoscenza del problema, frasi fatte e banalità, ritengo necessario ribadire anche in quest'Aula la necessità di affrontare una questione divenuta ormai emergenza e di farlo con la dovuta attenzione così come è stato fatto nella nostra mozione. La storia delle tre sorelle Mirabal, ripetuta più volte in quest'Aula questa mattina, in realtà ci ricorda un episodio di coraggio femminile, non soltanto della morte di donne, ma un atto di coraggio nel quale loro hanno difeso

Quindi, cacciamolo fuori anche noi tutto questo coraggio. Impariamo a diffidare da segnali che diventano sempre più chiari ed assillanti. Decidiamoci velocemente nel chiedere aiuto; facciamo sentire la nostra voce; riponiamo la fiducia nelle Forze dell'ordine. Sabato scorso ho incontrato alcune poliziotte che mi hanno raccontato della loro esperienza, anche difficile, da donna a donna, dinanzi ai fenomeni di *stalking* e di femminicidio ai quali lavoravano. Ebbene, solo il giorno prima si era rivolta a loro una giovane donna la quale ha riferito che sospettava che un'amica fosse oggetto di violenza da parte del marito (sempre in famiglia). È bastata una telefonata e la vittima le ha ringraziate. Ha detto che era felice di questa mano che le veniva finalmente tesa. Facciamo quindi appello appello anche a quella solidarietà femminile che troppe volte viene a mancare e che invece può essere il primo gradino verso quell'autonomia di pensiero che può spingere la vittima a chiedere aiuto. Ritengo superfluo, in questa sede, riportare conteggi, numeri e dati. In questi giorni ognuno di noi avrà avuto modo di leggerne tantissimi: fredde percentuali che poco raccontano se non attraverso il segno +, costante. Ognuno di noi, o per conoscenza diretta o per episodi accaduti nella propria comunità, sa bene quali segni profondi lascino tali crimini, soprattutto quelli delittuosi. In fondo, anche solo per un attimo, siamo tutti colpevoli. E allora è lì che dobbiamo agire e chiedere che gli uomini non siano più quelli che stanno a guardare le nostre manifestazioni ma che siano loro protagonisti di una difesa che ha la necessità di travalicare i limiti imposti da una società che noi non riconosciamo più. Non devono più sminuire gli allarmi lanciati dalle donne. Io sono stata oggetto di *stalking* per tre lunghi anni da parte di uno sconosciuto. È solo a ricordarlo vi assicuro che mi turbo. Mi sono sentita chiedere le cose più paradossali che mi facevano passare subito da vittima a inquisita, ma non è assurdo tutto questo? Un simile atteggiamento non limiterebbe chiunque nel denunciare, nel far valere i propri diritti, nel chiedere ragione di essere difesa e aiutata? Solo la mia insistenza ha fatto aprire le indagini. Ebbene, io sono stata fortunata ma non oso pensare a quelle donne che non hanno la mia capacità di persuasione. Ora, però, sia chiaro: le cose stanno cambiando. Il nostro Governo sta mettendo in essere una serie di interventi concreti a cominciare dai finanziamenti, dei quali si è parlato tanto e che tanti dicono che mancano ma finalmente ci sono,

Tutto questo in perfetta linea con la nostra mozione che si basa su 14 punti dei quali mi fa piacere sottolineare, in particolare, il valore dell'ultimo nel quale si Governo l'impegno a tutelare le donne, tutte le donne, nell'esercizio dei diritti e delle libertà loro riconosciute dalla nostra Costituzione e per garantire che l'effettiva condivisione dei valori in essa sanciti sia un requisito fondamentale per un reale processo di integrazione. Ebbene, il riferimento al profondo senso di equità della nostra Carta costituzionale rende ancora più apprezzabile la nostra mozione. Certo, sono i primi passi e bisognerà lavorare molto sulla cultura, sul rispetto e sul vero significato della parola «amore», «amore», ma la nostra mozione è un bel punto di partenza. Dichiaro quindi il voto favorevole del Gruppo del MoVimento 5 Stelle alla nostra mozione.

la premessa e il dispositivo - chiedo, anche conseguentemente al fatto che il Parlamento ha legittimamente scelto di non confluire su un unico testo ma di mantenere le posizioni originali, di votare per parti separate le premesse e i dispositivi.

Il Senato*,* in sede di esame del disegno di legge recante - Delega al Governo per l'adozione di disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi adottati in attuazione della delega per la riforma delle discipline

in attuazione della delega per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui alla legge 19 ottobre 2017, n. 155*** L'esigenza deriva dal fatto che la delega, di cui alla legge 19 ottobre 2017, n. 155, non ha previsto l'adozione dei decreti correttivi, la cui emanazione, nel contesto di una riforma complessiva della disciplina dell'insolvenza e della crisi di impresa, destinata ad avere un impatto rilevantissimo sull'intero sistema imprenditoriale e sull'operato degli uffici giudiziari interessati, si impone come assolutamente necessaria. Per l'esercizio della delega, da effettuarsi nel rispetto dei princìpi e dei criteri direttivi già fissati nella citata legge n. 155 del 2017, è prevista la fissazione di un termine di due anni, che decorre dalla scadenza del termine ultimo stabilito per l'acquisto di efficacia delle disposizioni dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega principale. L'individuazione di un tale *dies a quo* per l'esercizio della delega correttiva deriva dall'opportunità che sia previsto, nei decreti legislativi emanati in attuazione della delega principale, un ampio periodo di *vacatio,* analogamente a quanto stabilito in occasione delle riforme strutturali e di sistema, come quella sull'insolvenza e sulla crisi d'impresa. La proposta normativa è articolata in due disposizioni, la prima delle quali contiene la delega al Governo, mentre la seconda reca disposizioni finanziarie. Per recepire il parere della Commissione bilancio è stato successivamente approvato un emendamento che ha stabilito che, dall'attuazione delle disposizioni di cui l'articolo 1 della presente legge, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

legge, per il Partito Democratico emergono dubbi di due tipi. La prima perplessità concerne la natura stessa del provvedimento. La formulazione lascia infatti incerta la qualificazione tra una proroga dei termini precedenti e una delega nuova a tutti gli effetti. In entrambi i casi il Parlamento sarebbe comunque spettatore, dato che il testo consente di adottare disposizioni integrative e correttive nel rispetto dei princìpi e dei criteri direttivi fissati, però, dalla legge precedente. precedente. La seconda forzatura riguarda l'eccessiva ampiezza del periodo di *vacatio*: per l'esercizio della delega è fissato, infatti, un termine di due anni, che decorre però dalla scadenza del termine ultimo stabilito per l'acquisto di efficacia delle disposizioni dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega principale. Si tratta di un termine palesemente troppo lungo, come emerso già nel lavoro in Commissione, dove è stato respinto proprio l'emendamento Caliendo, che dimezza il termine, con un parere non ostativo - mi riferisco alla Commissione affari costituzionali - nel presupposto, però, che il disegno di legge sia approvato, in via definitiva, successivamente all'adozione di almeno uno dei decreti legislativi in attuazione della delega di cui alla legge n. 155

noi diremo no al provvedimento in esame, anche per via di un atteggiamento di questo Governo, che pare nutrirsi troppo spesso di incostituzionalità e noi speriamo che ne faccia indigestione. *(Applausi

ci sembra un po' troppo, tenuto conto che gli ambienti forensi - e non solo - e tutti coloro che sono interessati a

di una liquidazione giudiziale in cui si accompagna chi è in crisi, attraverso l'istituto dell'allerta,

professionisti che possono intervenire, sia al sovraindebitamento, che dev'essere considerato in maniera specifica. Le audizioni svolte ci hanno dato un gran conforto. Mi auguro che, nell'esprimere il proprio parere, la Commissione giustizia del Senato tenga conto di tali necessità e che il Governo poi, nell'emanare il decreto-legge definitivo,

In pratica, la legge prevedeva che il Governo, attraverso i decreti attuativi, formulasse una sostanza del codice del fallimento che mettesse ordine nella variegata materia che fino ad oggi ha regolato la crisi d'impresa.

l'ordinamento concorsuale italiano alle direttive europee, che imponevano l'adozione di procedure di composizione nelle crisi d'impresa fondate essenzialmente sul criterio della prevenzione della continuità aziendale. A questo ci si era attenuti, quando, nella scorsa legislatura, era stata approvata la legge delega. Oggi si porta all'esame del Parlamento un testo che sostanzialmente è un monoarticolo, oltre alla clausola d'invarianza finanziaria, nel quale di fatto si riapre tutta la materia. Perché dico questo? I decreti attuativi non erano stati emanati: come dicevo, la delega scadeva il 17 novembre 2018 e, di fatto,

per il decreto attuativo i rami del Parlamento sono chiamati a dare il loro parere e, quindi, a formulare tutte le osservazioni necessarie, che sicuramente sono da fare anche in maniera critica su alcuni aspetti.

Non è una proroga, perché, se fosse stata tale, avremmo detto semplicemente che i termini stabiliti vengono prorogati di un certo lasso di tempo. No: qui si dà una delega che è molto più vasta e che di fatto consentirà al Governo di spazzare via tutto e di riscrivere tutto.

Signor Presidente, il nostro Gruppo su questo provvedimento si asterrà, perché lo leggiamo come una sorta di delega in bianco su una materia estremamente delicata,

Paese. Quando si dice che si vogliono tutelare i poveri, questi ultimi devono trovare una soluzione in questo schema di decreto, perché i poveri sono quelli che hanno avuto la casa pignorata a seguito di una fideiussione mal posta; i tutti coloro che hanno subìto le conseguenze di una crisi che dura da dieci anni. Sono i professionisti, anche loro interessati a questo tipo di problematica; sono le imprese, che sono saltate per aria e non riescono ad avere soluzioni sulla base della normativa. Questo provvedimento è il cuore Il Governo aveva fatto delle scelte. La maggioranza, quando ha voluto compiere un salto con riferimento - ad esempio - alla delega sull'ordinamento penitenziario, ha fatto delle proroghe per altri, ma ha agito dando

abbiamo una delega in bianco; preghiamo i Gruppi, anche e soprattutto quelli di maggioranza, di esaminare con attenzione

esclusivamente della possibilità che Parlamento e Governo devono avere di apportare eventuali correttivi a una delega. Ma il dispositivo - lo cito testualmente - reca «nel rispetto dei principi e criteri direttivi» fissati dalla legge n. 155 del 2017, cioè dalla legge delega istitutiva. Non c'è, quindi, una volontà

ispettivo. *(La seduta, sospesa

in quanto vertono su analogo argomento. In via generale, occorre premettere che la Direzione generale per il trasporto stradale e l'intermodalità del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti autorizza l'esercizio di servizi di linea di competenza statale per il trasporto di passeggeri con autobus che attraversano più di tre Regioni, servizi internazionali comunitari e servizi internazionali con Paesi extra Unione europea. europea. Le aree di fermata per i predetti servizi sono individuate esclusivamente dall'ente proprietario della strada, nella fattispecie Roma capitale. Perché possano essere utilizzate, lo stesso ente deve provvedere alla richiesta del nulla osta alla sicurezza, che viene rilasciato dall'ufficio di motorizzazione civile territorialmente competente, solo all'esito degli interventi di approntamento dell'area. Attualmente a Roma sono attive solo due aree di fermata per gli autobus di competenza statale, l'autostazione Tiburtina e la fermata di Anagnina. Tuttavia pressoché tutti i servizi di linea utilizzano la prima, in quanto semicentrale, dotata di migliore connessione modale (treno e metropolitana) e costantemente presidiata. Tutto ciò premesso, sulla questione in argomento il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha espresso, come in reiterata corrispondenza con il Comune di Roma, tutte le proprie perplessità in ordine allo spostamento dell'autostazione da Tiburtina (come detto semicentrale e dotata di buone connessioni modali) ad Anagnina, lontana dal centro e priva di collegamento con il trasporto ferroviario. Tali perplessità nascono quindi dall'ubicazione decentrata della nuova autostazione, da una minore integrazione modale, da problemi di sicurezza dei viaggiatori, specie nelle ore serali e notturne, oltre che dalla dubbia adeguatezza dei servizi e degli spazi rispetto al flusso di veicoli e persone ne deriverebbe. Il Ministero però, pur essendo a conoscenza dell'ipotesi di spostamento e pur ritenendola fortemente penalizzante, non ha alcuna possibilità di intervento, considerato che, come premesso, la localizzazione dell'area di fermata è di esclusiva competenza dell'ente proprietario della strada. Tuttavia, continuerà a prestare ascolto alle notevoli segnalazioni che pervengono da associazioni di settore, utenti e imprese, nell'auspicio di poter trovare una soluzione adeguata e condivisa con Roma capitale. Signor Presidente, per la verità mi ritengo insoddisfatto della risposta del Governo, anche se il Governo ammette

dall'Abruzzo e dalle Marche) sia penalizzante per tutta l'utenza e per i tanti viaggiatori che sono costretti a recarsi in pullman a Roma, riconoscendo che questo spostamento da Tiburtina ad Anagnina provocherebbe un danno enorme, anche collegato al problema dell'intermodalità dato che quando si arriva a Tiburtina c'è la possibilità di prendere anche il treno e non solo i mezzi urbani o la metropolitana. Appare infatti evidente che questa è una risposta

di pendolari provenienti da Regioni italiane, che già sono sottoposti a un trattamento particolarmente penalizzante (quello di recarsi per motivi di lavoro

e nelle Marche - ovviamente, essendo abruzzese, parlo innanzitutto per gli abruzzesi - non hanno possibilità alternative di recarsi a Roma.

linee ferroviarie da Medioevo. Gli spostamenti pertanto necessariamente sono a mezzo autobus, che percorre l'Autostrada dei Parchi, di cui tanto si è parlato ultimamente. Avendo

la ragione per la quale noi riteniamo che sia assolutamente necessario che il Governo si impegni affinché si impedisca un trattamento così penalizzante nei confronti

Essa verte sulla decisione della Giunta Raggi del Comune di Roma di spostare dalla sede della Tiburtina una stazione degli autobus che è di livello non solo interregionale,

una sciagura che impatterà sulla vita quotidiana e concreta di migliaia di persone. La buona amministrazione significa prendersi cura; invece, è uno schiaffo in faccia. Lei sa, Sottosegretario, che sono 8 milioni ogni anno le persone che usufruiscono di quell'*hub* internazionale, ogni giorno più di 18.000.

per arrivare a Roma e la sera rientrare a casa. Sono molto spesso studenti fuori sede. Infatti, attorno al quartiere della Tiburtina vi sono le abitazioni della gran parte degli 80.000 studenti fuori sede delle università romane. Utilizzano quegli autobus, perché è un vero e proprio servizio pubblico, coloro che non possono permettersi di utilizzare i mezzi privati, le automobili o i treni, quindi le persone più deboli. La Tiburtina,

tra la periferia e il centro; questa scelta contribuirà a un ulteriore strappo. Servono, invece, idee e progetti. Se vi è un problema di concessione, si risolva, si utilizzino soldi non per Anagnina, ma per riqualificare Tiburtina, che è davvero una scelta strategica. Sottosegretario e Governo, state dalla parte dei cittadini italiani e dei romani, non dalla parte della sindaca Raggi, e fermate questo scempio.

l'Abruzzo, le Marche, il Molise, tutta la provincia romana, in particolare quella Est che corre lungo gli assi tiburtino, nomentano, casilino, che finiscono appunto verso la stazione Tiburtina, dove arrivano i pendolari che si svegliano alle quattro mattina per essere puntuali a Roma nei loro uffici o nelle aule universitarie. Infatti, vicino alla stazione Tiburtina c'è il più grande ateneo d'Europa, con decine di migliaia di studenti fuori sede che la mattina fanno pendolarismo per arrivare lì e che, con la decisione di essere spostati su Anagnina, peggiorata la loro qualità della vita, perché impiegherebbero almeno altri trenta o quaranta minuti di viaggio solo per prendere la metropolitana e raggiungere l'estrema periferia, dove oggi è collocata

più lungo di almeno 3 chilometri. Inoltre, se moltiplichiamo questi 3 chilometri dell'andata con quelli del ritorno per centinaia di *pullman* al giorno per tutto l'anno, arriviamo a milioni di chilometri/vettura, di scarichi, di inquinamento, di tempo perso, di peggioramento della qualità della vita per i romani,

sicuramente bene a farlo e vogliamo sperare che la vostra azione volta a farle capire che deve tornare indietro possa portare a un risultato. Tuttavia, il Ministero ha delle precise competenze perché, per autorizzare

e quando capisce che questi criteri non sono garantiti, il Ministero deve intervenire in maniera perentoria nei confronti dell'amministrazione comunale e impedire una scelta stupida e sbagliata di un'amministrazione

intende adottare per dare risposta adeguata alle istanze dei ricercatori precari, si precisa quanto segue. In via preliminare occorre evidenziare che, a monte della questione in esame, esiste una sostanziale differenza di intenti tra le legittime aspettative del personale addetto alla ricerca presso gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) di diritto pubblico e di quelli in servizio presso gli istituti zooprofilattici sperimentali

Infatti, a fronte della richiesta di una stabilizzazione a posto fisso, non viene seguito un *iter* legato alla produttività, bensì un percorso che prevede l'emanazione di appositi bandi di concorso per il personale della ricerca titolare di contratto a tempo determinato, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 75 del 2017. La differenza di regime deriva dal differente modo di finanziamento delle linee di ricerca, che in taluni casi viene attuato tramite l'erogazione di importi fissi e predeterminati, mentre, nel caso della ricerca corrente e finalizzata, varia di anno in anno, a seconda degli obiettivi prefissati ed effettivamente conseguiti dalle differenti realtà degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico Più in particolare, in merito alla disciplina attualmente vigente e alle iniziative poste in essere per la sua puntuale e compiuta attuazione, nonché al funzionamento e agli obiettivi della cosiddetta piramide dei ricercatori, di cui all'articolo 1, commi 422 - 434, della legge del 27 dicembre

rinnovabile per ulteriori cinque anni, con la possibilità, una volta completato positivamente il secondo periodo del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, di inquadramento a tempo indeterminato nei ruoli del servizio sanitario nazionale.

La normativa introdotta dalla legge n. 205 del 2017 persegue l'obiettivo di intervenire in modo organico sul personale della ricerca sanitaria, nell'ottica di salvaguardare la continuità di carriera del ricercatore e nel rispetto della flessibilità tipica nel contesto della ricerca e del principio della competitività, in piena sintonia con il sistema altamente concorrenziale in cui agiscono gli enti di ricerca sanitaria. Per quanto riguarda i ricercatori già in servizio, la legge n. 205 del 2017 dispone all'articolo 1, comma 432, una specifica disciplina che prevede l'accesso al predetto percorso per il personale in possesso dei requisiti previsti dalla normativa e, quindi, in servizio presso gli IRCCS e gli istituti zooprofilattici sperimentali (IZS) al 31 dicembre 2017, con rapporti di lavoro flessibili instaurati a seguito di procedura selettiva e con un'anzianità di servizio di almeno tre anni negli ultimi cinque. Al fine di conferire un riconoscimento professionale allo *status* dei ricercatori è stato istituito il ruolo della ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla stessa

Quanto alla procedura per l'emanazione dei decreti attuativi della normativa in questione, si segnala che è stato predisposto uno schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per la disciplina concorsuale e sono stati costituiti due gruppi di lavoro, uno per i ricercatori e uno per il personale di supporto, ai fini della definizione dei criteri di valutazione annuale

quesito che avevo rivolto riguardava il fatto che la gran parte di questi ricercatori è in scadenza il 31 dicembre 2018. Attualmente molti di questi, dopo anche venti anni di lavoro, rischiano di dover interrompere il rapporto di lavoro con l'IRCCS e attualmente gli istituti si stanno in sostanza arrangiando da soli. chi rischia di interrompere il rapporto di lavoro, lasciando quindi senza lavoro queste persone e c'è chi, invece, autonomamente, ha deciso di riaprire altri concorsi in modo da salvaguardare un patrimonio prezioso per l'istituto e per l'intera sanità pubblica.

Altri di questi ricercatori lavorano da molti anni con borse di studio e nulla è previsto in questo momento per il futuro di queste persone.

sanità, mentre i medici, i biologi e i chimici sono inquadrati nella dirigenza del Servizio sanitario nazionale. È questo un ulteriore fattore di demotivazione, che renderebbe poco attrattivo questo lavoro, altrimenti preziosissimo Sottosegretario Bartolazzi, acquisiremo la risposta, che mi viene detto essere più lunga, agli atti, in maniera tale che la senatrice potrà prenderne visione.

Signor Presidente, onorevoli senatori, prima di entrare nel merito delle questioni poste con l'atto di sindacato ispettivo, occorre premettere che Matera - sito riconosciuto patrimonio universale dell'umanità da parte dell'UNESCO sin dal 1993 ha effettivamente visto aumentare in maniera esponenziale il flusso turistico a seguito della designazione della città, avvenuta il 17 ottobre 2014, a capitale europea della cultura per il 2019. Al conseguente, significativo aumento delle presenze turistiche dal 2014, ha fatto seguito un corrispondente incremento di attività commerciali, soprattutto nell'ambito della ristorazione e delle strutture ricettive, sia all'interno del rione dei Sassi che nel resto del capoluogo. Peraltro, l'unicità dei luoghi in questione e l'eco mediatica che sarà conseguente alle iniziative del prossimo anno fanno ritenere che l'attrattività turistica del sito non diminuirà anche in futuro. Tanto premesso, si rappresenta che la questione dell'esigenza di riclassificare, da un lato, e di potenziare temporaneamente, dall'altro, l'organico del personale operativo del comando provinciale dei Vigili del fuoco di Matera è oggetto di massima attenzione da parte del Ministero dell'interno. Infatti, sebbene il predetto comando conti attualmente la presenza di 191 unità di personale operativo a fronte di una dotazione teorica di 182, l'accresciuto carico antropico e di attività commerciali, non disgiunto dalla difficoltà di raggiungimento dei locali nei cosiddetti Sassi (la gran parte dei quali si sviluppano quasi in verticale per diversi metri sottoterra) e le particolari caratteristiche della viabilità della zona, suggeriscono un'attenta valutazione della situazione. A tal proposito, si riferisce che è allo studio una soluzione per il temporaneo potenziamento dell'organico, misura che permetterebbe al comando di Matera di avere sempre la disponibilità di almeno due squadre operative. Inoltre, si sta valutando di garantire un presidio giornaliero dinamico costituito da una squadra dedicata alle iniziative legate a Matera 2019, dislocata all'interno della zona dei Sassi, in servizio diurno straordinario durante tutto l'anno 2019. Il presidio assumerebbe carattere dinamico in quanto, vista la difficoltà di raggiungere il centro storico, caratterizzato da eccezionale affollamento in presenza di particolari manifestazioni, si prevede la presenza sul posto, in regime di lavoro straordinario, di personale con professionalità e abilitazioni diversificate (quali quelle di primo soccorso sanitario, le Speleo-Alpino-Fluviali, le telecomunicazioni), in modo da poter garantire interventi di varia tipologia, ma modulabili in funzione dell'impegno reale richiesto dalle caratteristiche del singolo evento. Il presidio avrebbe, quindi, modalità di impiego flessibili e come base logistica alcuni locali messi a disposizione dall'amministrazione provinciale, ove saranno ricoverati anche mezzi ed attrezzature di servizio. Attualmente, in particolare per l'attivazione del predetto presidio dinamico, sono in fase avanzata ì contatti con la Regione Basilicata, tenuti tramite la prefettura di Potenza, al fine di pervenire alla stipula di un'apposita convenzione per concorrere alla copertura dei connessi oneri economici. Nell'avviarmi alla conclusione, mi preme anche evidenziare come il Governo sia, più in generale, fermamente deciso a potenziare la capacità operativa del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco attraverso un consistente rafforzamento degli organici. Infatti, nel disegno di legge di bilancio per il 2019, che è attualmente all'esame di questo ramo del Parlamento, abbiamo previsto, nell'ambito di un più ampio piano straordinario, l'assunzione di 1.500 Vigili del fuoco secondo la seguente tempistica: 650 unità dal 10 maggio 2019, 200 unità dal 1° settembre 2019 e 650 unità dal 1° aprile 2020. Si tratta di un primo concreto e importante risultato di un'azione che il Governo intende sostenere e ampliare con assoluta determinazione a beneficio di un comparto da sempre a servizio dell'incolumità e della sicurezza dei cittadini.

e del sottodimensionamento degli organici che affligge un po' tutte le Forze dell'ordine italiane e le Forze di sicurezza. Quella di Matera è una vicenda che ha già visto dei problemi all'interno del rione Sassi in occasione di eventi calamitosi molto recenti. Quindi, preoccupa tutta la nostra comunità che lo sviluppo impetuoso del turismo e delle attività ricettive che stiamo registrando in questi anni non sia accompagnato da una attenzione della pubblica amministrazione. Registriamo con favore gli impegni del Governo per potenziare il comando provinciale e istituire questo temporaneo potenziamento dell'organico, a cui siamo certi farà seguito una sistemazione più stabile. Pertanto, salutiamo con favore l'intervento che il Governo vorrà fare per la città dei Sassi, per Matera, per la Basilicata e per il prestigio internazionale che il prossimo appuntamento darà a tutta l'Italia.

efficacemente l'odioso fenomeno delle violenze verbali espresse in rete, anche favorendo l'*iter* di disegni di legge relativi all'istituto della diffamazione, che estendano le disposizioni di cui all'articolo 595, comma 3, del codice penale in materia di diffamazione a mezzo stampa, alle offese, agli insulti ed alle affermazioni particolarmente lesive della dignità della persona, genericamente diffuse ed inneggianti a qualunque forma di violenza. Ed ancora, se non ritenga, nei casi in cui le violenze verbali siano rivolte in danno del genere femminile, promuove iniziative volte a prevedere delle aggravanti speciali di pena, anche alla luce dei sempre più diffusi tragici casi di femminicidio, divenuti ormai un'emergenza nel nostro Paese.

Cito: «Piddine, fatevi stuprare dagli immigrati. Allora è come dice il mediatore culturale idiota, all'inizio fa male; poi, buon divertimento». A ciò seguivano ulteriori commenti sessisti e lesivi della dignità femminile, che inducevano la dottoressa Gasparini a presentare querela per i reati di istigazione a delinquere, diffamazione e minaccia. Nel merito della specifica vicenda richiamata nell'atto di sindacato ispettivo, il Ministero ha provveduto ad acquisire elementi conoscitivi presso gli uffici giudiziari titolari del relativo fascicolo, che confermano quanto riportato nell'atto di sindacato ispettivo. In particolare, a seguito della querela presentata dalla dottoressa Gasparini l'8 settembre 2017, la procura della Repubblica di Modena apriva un procedimento, rubricato al n. 7404/17 RG NR Mod.21 a carico del sopracitato Montorsi ed altri, per i reati di istigazione a delinquere, diffamazione e minaccia di cui agli articoli 414, 595 e 612 del codice penale, che veniva definito dal pubblico ministero titolare delle indagini in data 13 ottobre 2017 con richiesta di archiviazione per insussistenza del fatto. In accoglimento di tale richiesta, cui seguiva l'opposizione della parte offesa, il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Modena, con decreto del 2 luglio 2017, disponeva l'archiviazione del procedimento. Va preliminarmente osservato che, rispetto alla decisione assunta nella fattispecie concreta, esula dalle prerogative del Ministro della giustizia esprimere ogni tipo di valutazione in ordine al merito dei provvedimenti assunti dall'autorità giurisdizionale, così come è riservata in via esclusiva all'autorità giudiziaria l'attività di interpretazione delle norme di diritto. Ciò premesso, con specifico riguardo all'invocata estensione delle disposizioni di cui all'articolo 595, terzo comma del codice penale: «anche alle offese, agli insulti e alle affermazioni particolarmente lesive della dignità della persona» comprese quelle «genericamente diffuse e inneggianti a qualunque forma di violenza», non è dato riscontrare nel nostro ordinamento un vuoto normativo di tutela penale. L'attuale assetto normativo è, infatti, già astrattamente idoneo a punire pure tali condotte, purché risulti individuabile la persona la cui reputazione possa reputarsi lesa. In particolare, secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza della Suprema Corte, e recepito da quella di merito, il reato di diffamazione è costituito dall'offesa alla reputazione di una persona determinata e non può essere, quindi, ravvisato nel caso in cui vengano pronunciate o scritte frasi offensive nei confronti di una o più persone appartenenti ad una categoria anche limitata se le persone cui le frasi si riferiscono non sono individuabili. Per il configurarsi di una diffamazione a mezzo stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, deve sussistere la lesione della reputazione altrui (sia essa persona fisica, giuridica, partito, gruppo, comitato, associazione), purché il soggetto offeso sia almeno individuabile. Pertanto, tale delitto può senz'altro integrarsi anche in caso di offesa alla reputazione di un partito politico. In tal senso è stato, infatti, deciso che in tema di diffamazione a mezzo stampa, se si reca offesa alla reputazione di un partito politico, attraverso il comportamento attribuito a suoi esponenti non identificati, che agiscono in un determinato territorio, legittimato a proporre querela è chi legalmente lo rappresenta in quel territorio.

per arrivare ad avere, anche da questo punto di vista, delle sanzioni. Lo so che è difficile perché individuare l'attore, individuare chi ha commesso l'istigazione all'odio sui *social network* è sicuramente difficile però io credo che si debba integrare, ormai, come si sta facendo in tutto il mondo, il nostro sistema penale.

in raccordo con gli organi locali competenti.

Allo stato, pertanto, oltre la sede circondariale a integrale gestione statale, sono previsti gli uffici del giudice di pace di Casarano, Gallipoli, Tricase e Ugento che operano secondo l'assetto e la funzionalità delle sedi mantenute, ai sensi del suddetto decreto legislativo n. 156 del 2012, secondo cui le spese di erogazione del servizio giudiziario, ivi incluse quelle inerenti al

infatti, che, qualora l'ente locale responsabile della gestione del presidio giudiziario non rispetti gli impegni relativi al personale amministrativo ed alle spese per un periodo superiore ad un anno, il relativo ufficio del giudice di pace sia soppresso mediante l'adozione di un decreto ministeriale che provvede all'esclusione

rilevanza, se posto a confronto con quello relativo al limitrofo distretto di Taranto, ove, a fronte di una pianta organica di 465 unità, risultano coperti 383 posti, tenuto conto anche delle posizioni di distacco e comando, con una percentuale di scopertura media del 17,63 per cento o a quello dell'altrettanto contiguo distretto di Bari, ove, rispetto ad una pianta organica di 1.520 unità, risultano coperti 1.312 posti, 1.312 posti, tenuto conto anche delle posizioni di distacco e comando, con una percentuale di scopertura media del 13,68 per cento. Più specificatamente, con riferimento al distretto di Lecce si osserva che, quanto al personale con qualifica di assistente giudiziario,

altri 200 assistenti giudiziari, mediante ulteriore scorrimento della graduatoria del concorso. Al riguardo si rappresenta altresì che, con decreto ministeriale 14 febbraio 2018, l'amministrazione ha già modificato la dotazione organica del profilo

formali proposte in tal senso. Al momento a Moena è operativo un comando stazione dell'Arma dei carabinieri, oltre a un comando della polizia locale. Peraltro, dall'esame dei relativi dati, si evince una sensibile riduzione, pari al 19,7 per cento, della delittuosità nel predetto Comune nel periodo gennaio-ottobre 2018, se In merito alle preoccupazioni sollevate dall'interrogante circa i disagi patiti dai cittadini relativamente alla necessità di recarsi a Trento per il disbrigo delle pratiche amministrative, faccio presente che - come accade peraltro per altre aree posizionate nelle valli del Trentino, presso il Centro addestramento alpino della Polizia di Stato di Moena è stato già appositamente organizzato ed operante uno "sportello periferico" portatile con l'intervento di personale della questura di Trento che, una volta al mese, garantisce la propria presenza sul territorio per agevolare l'acquisizione e la consegna dei passaporti e dei documenti di accompagno per i minori di quindici Se allo stato, pertanto, non sembrano sussistere i presupposti per l'istituzione di un posto fisso di polizia a Moena, posso assicurare, in linea più generale, che alta è l'attenzione di questo Governo sull'esigenza di garantire al territorio della Provincia di Trento più alti *standard* di sicurezza. Da questo punto di vista informo che è già in corso l'attuazione, da parte del Ministero dell'interno, di un apposito piano di potenziamento degli organici di tutte le questure, nell'ambito del quale è stata già programmata l'assegnazione a Trento di complessive 21 unità di personale, delle quali 12 già assegnate ad ottobre scorso, un'unità da assegnare entro il prossimo mese di dicembre al Centro di addestramento di Moena e altre 8 a decorrere dal mese di febbraio 2019. Intendo ribadire, anche in questa occasione, l'intenzione del Governo di innalzare l'efficacia dell'azione di prevenzione e contrasto delle Forze di polizia, migliorando ulteriormente gli *standard* di operatività del sistema sicurezza. In tale direzione si iscrive lo stanziamento di 500 milioni di euro nel disegno di legge di bilancio per l'anno 2019,

Stato, che erano state ridotte a 106.000 unità dalla legge Madia e, intanto, non abbiamo dato seguito al progetto di riduzione dei presidi di sicurezza in tutto il Paese, che era stato proposto dal Governo precedente, perché siamo convinti che occorra salvaguardare le specificità della Polizia, potenziandone gli assetti e non riducendoli.

Vorrei sottolineare l'importanza del Centro addestramento alpino di Moena, che nasce nel 1948 da un primo corso di addestramento per sciatori tenuto dagli alpini, poi è stato spostato nel 1952 proprio a Moena, in una località turistica di grande rilevanza che è la Valle di Fassa. Qui si è costruita da sempre una formazione per il personale addetto alla sicurezza e al soccorso di montagna,

dunque utilizzato per aiutare tutte le persone che vivono le difficoltà della montagna. Questa struttura da anni non ospita più corsi per allievi, salvo un corso semestrale di base riservato alle Fiamme oro, in fase sperimentale. Si tratta quindi di una struttura che viene

di spopolamento, che può essere contrastato solo ed esclusivamente mantenendo i servizi per i cittadini che vivono la montagna. Su questo punto vorrei insistere, proprio perché, se non si garantiscono i servizi ai territori non urbani, voglio capire come si può contrastare

alle quali risponderanno il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e il Ministro per i beni e le attività culturali. Invito gli oratori ad un rigoroso rispetto dei tempi, considerata la diretta televisiva in corso. Il senatore Casini

il primo Paese a riaprire l'ambasciata a Tripoli. Questo va a onore dell'Italia e della nostra diplomazia. Apro una parentesi e la chiudo: dal segretario generale all'ultimo funzionario, possiamo essere fieri dei nostri diplomatici, che, indipendentemente dai Governi che si susseguono, fanno un lavoro serio nell'interesse del Paese. Dobbiamo essere particolarmente grati a quanti operano in condizioni difficili, come in Venezuela o, nel caso dell'interrogazione, in Libia. Si dà il caso, però, che dal 20 agosto, noi, che pure abbiamo abbiamo intrapreso un'iniziativa a Palermo, due settimane fa, nella Conferenza sulla Libia, abbiamo una sede priva dell'ambasciatore, il quale ha fatto un'intervista successivamente è stato invitato a rientrare (ma non si capisce in base a quali ragioni, veramente). Ieri ho esaminato i testi delle sue risposte in Commissione affari

tutta la preparazione della vicenda della Conferenza per la Libia ha visto assente uno dei suoi principali conoscitori e soprattutto nostro ambasciatore in Libia. È come se facessimo una Conferenza su un altro Paese senza il nostro ambasciatore, che

anche diverse. Vorrei dunque che si definisse con chiarezza la ragione per cui l'ambasciatore è qui. Se non può rientrare, nominatene un altro e destinate questa persona - che, peraltro, è un profondo conoscitore del mondo arabo - a fare qualche cos'altro; se il nostro

Vorrei anche chiarire che l'ambasciatore Perrone è stato fatto rientrare in Italia, Roma, il 10 agosto e da allora non ha fatto ritorno in Libia. La decisione, presa

Su questo punto ho avuto modo di riferire anche in Aula e mi duole se non sono stato sufficientemente bravo ad esprimermi con chiarezza, ma spero di essere chiaro in quest'occasione. Il Governo intende assicurare la presenza del capo missione a Tripoli nei tempi

la questione della presenza di un capo missione come urgente, non più differibile e da risolvere nei tempi più rapidi. Il Governo sta già facendo tutte le opportune valutazioni al fine di assumere quanto prima questa decisione.

voglio far finta che sia mezzo pieno. La ringrazio del fatto che lei, dopo cinque mesi, conviene con me sul fatto che sia indifferibile la nomina di un altro ambasciatore, visto che non c'è l'agibilità per questo in Libia. A questo punto aspetto la nomina e sicuramente, conoscendola e stimandola, so che sarà una nomina all'altezza della situazione. Solo alla fine, per quel po' di polemica che un pochino ciascuno di noi mette, accaduto era dovuto alla sicurezza dell'ambasciatore o al fatto che autorità anche italiane operanti in Libia hanno idee diverse rispetto alla valutazione che l'ambasciatore faceva in ordine alla situazione libica. Parlano tutti di Libia: le autorità di sicurezza, i Servizi, il Ministero degli esteri. C'è molta confusione e duplicazione di competenza. Io credo che i Servizi che agiscono in Libia,

entrato in un meccanismo più grande di lui, per cui alla fine abbiamo sacrificato l'ambasciatore. Benissimo, adesso comunque nominiamone un altro e guardiamo avanti, non guardiamo più indietro; stendiamo un velo sul passato. Come lei ha detto - e io sono d'accordo con lei - bisogna rapidamente provvedere all'indicazione di un altro ambasciatore. **Saluto

Signor Presidente, onorevole Ministro, il 10 e 11 dicembre si terrà a Marrakech la Conferenza intergovernativa per l'adozione del Global compact, il patto globale sull'immigrazione. Per Fratelli d'Italia questo patto farà cadere ogni distinzione tra chi è profugo,

Contro questo approccio immigrazionista e a favore invece della sovranità nazionale si sono già schierati gli Stati Uniti, il gruppo di Visegrád (Ungheria, Polonia, Repubblica Ceca e Slovacchia), nonché l'Australia, l'Austria

che sancisce di fatto la migrazione come un diritto universale e incontrollato. E per il nostro Paese, per la sua centralità nel Mediterraneo, per la sua centralità nel continente liquido che è il Mediterraneo, questo aspetto è importantissimo, perché il nostro Paese rappresenta l'approdo delle rotte che provengono dall'Africa ed è anche la porta di accesso al mondo occidentale. tale patto per il nostro Paese è di un'importanza cruciale. Mi scuso se quanto abbiamo presentato differisce un po' da quello che dico, ma lei converrà con me, signor Ministro, che si sono registrati molteplici colpi di scena negli ultimi giorni e nelle ultime ore su questo tema. Sul Global compact si sono registrate dichiarazioni contrastanti e contraddittorie. Inizialmente, sia lei, signor Ministro, che il *premier* Conte avete espresso un orientamento favorevole alla sottoscrizione; poi, dopo giorni di silenzio, noi di Fratelli d'Italia abbiamo sollecitato una dichiarazione da parte del Governo; il ministro Salvini ha rinviato la decisione al parlamento ed il *premier* Conte ha dichiarato che l'Italia non parteciperà alla Conferenza di Marrakech. Allora, qual è, e se c'è, una posizione del Governo? Perché avete atteso tanto? Perché avete atteso fino all'ultimo minuto? Certo, non era una sorpresa la sottoscrizione del Global compact. Quali elementi ritiene di poter fornire a quest'Assemblea oggi rispetto a quella che è sembrata una marcia indietro dettata dalla paura di spaccare una compagine governativa dalla doppia anima, scegliendo quella del Parlamento come una via di fuga?

di qualunque questione, inclusa questa del cosiddetto Global compact for migration, quindi di questo patto per le migrazioni a livello multilaterale. Ero disponibile anche prima, qualora le Commissioni lo avessero richiesto.

non è neanche definibile «accordo» - che riguarda la migrazione sicura, ordinata e regolare, secondo il titolo che gli viene dato in lingua italiana, e rappresenta una piattaforma di cooperazione tra i Paesi partecipanti per governare i flussi migratori a livello internazionale, secondo un approccio multidimensionale di condivisione degli oneri tra i Paesi di origine, di transito e di destinazione dei migranti stessi. Questo per fornire un cenno di merito su cosa stiamo parlando, magari anche a beneficio dei ragazzi che stanno assistendo alla nostra seduta. mese per essere più precisi, avevo detto che avremmo avuto un approfondimento in sede di Governo: lo avevo detto in quest'Aula rispondendo a un'altra interrogazione parlamentare. Questo approfondimento in sede di Governo sarebbe dovuto avvenire - ed è poi avvenuto - prima di procedere alla conclusione eventuale, sottolineavo - del Global compact. E avevo aggiunto che avremmo tenuto conto anche degli stimoli parlamentari. In tal senso, successivamente ho scritto anche al Presidente del Consiglio per renderlo edotto di si era detto in quest'Aula. Questa posizione è stata confermata sostanzialmente ieri. In considerazione del fatto che il Global compact è un documento con una sua complessità, che tocca temi questioni estremamente sensibili e sentite dai cittadini, il Presidente del Consiglio ha comunicato che il Governo, dopo l'approfondimento, ritiene opportuno che ci sia un un dettagliato e articolato dibattito in Parlamento, a monte delle decisioni circa la scelta definitiva da fare. Sempre il Presidente del Consiglio ha avuto modo di precisare ieri che il Governo non parteciperà alla Conferenza, quindi nessun membro di Governo sarà presente alla Conferenza di Marrakech; l'Italia sarà rappresentata e il nostro Paese, sulla base degli esiti del dibattito parlamentare e dell'orientamento che a quel punto il Governo prenderà, potrà eventualmente in seguito valutare le scelte definitive da fare. Una posizione analoga la riscontriamo nella Confederazione Elvetica, o Svizzera che dir si voglia. *(Applausi dai Signor Ministro, grazie anche per i cenni di merito, ma in quest'Aula credo che li conoscessimo già tutti. Non ho trovato nelle sue parole, però, quale sia la sua posizione personale. Conosco quella che lei aveva espresso

in via definitiva ogni politica di contrasto all'immigrazione incontrollata per la mancata distinzione tra profughi e clandestini. Riteniamo che il fatto che il ministro dell'interno Salvini abbia delegato al Parlamento, chiedendo di agire secondo coscienza,

che il Global compact immigration sia contro l'interesse nazionale, non governi l'immigrazione, ma anzi la incoraggi in modo incontrollato, non sappia distinguere tra regolari e clandestini, minacci i confini e la sovranità e, soprattutto, abbia già fatto esplodere contraddizioni all'interno del Governo. È evidente che c'è un'anima mondialista e una sovranista che su questo punto non riescono a trovare un accordo, come non l'hanno trovato ieri al Parlamento europeo quando, votando su questo punto, i grillini, da un lato, e la Lega, dall'altro, si sono spaccati. Rimettere la decisione al Parlamento ci continua a sembrare anche oggi, dopo le sue parole, un atteggiamento pilatesco

*(PD)*. Ministro Centinaio, con la legge di bilancio per l'anno 2018, abbiamo introdotto la disciplina dell'attività di enoturismo, annunciata *in nuce* nel testo unico del vino e poi ripresa dall'attività parlamentare. La norma, come da prassi, contiene un espresso rinvio ad un apposito decreto interministeriale, da adottarsi d'intesa con la Conferenza per i rapporti tra Stato e Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, per delineare le linee guida definitive attuative. Ebbene, questo decreto c'è. È stato trattato nella riunione della Conferenza del 10 maggio scorso, dove il presidente Bonaccini, in nome delle Regioni, esprimeva avviso favorevole all'intesa, condizionandola all'accoglimento di minime proposte di modifica. Il vice ministro uscente di allora, Olivero, per cortesia istituzionale, ha proceduto al rinvio in attesa del nuovo Governo. Da qui non è accaduto più nulla. Mi sia permesso un breve inciso: il riconoscimento dell'enoturismo è il risultato di un'intensa attività istituzionale, di collaborazione e ascolto con tutta la categoria, che chiedeva una legittimazione normativa ad un *business* che vale almeno 3 miliardi all'anno e che muove già 15 milioni di turisti. La sua più volte dichiarata sensibilità riguardo al mondo del vino e del turismo, Ministro, lo dico con cortesia istituzionale, ha avuto negli ultimi mesi qualche in un'intervista del luglio scorso lei rimandava ad una condivisione immediata con le Regioni per le ultime limature, mentre qualche giorno fa era a Verona - poco prima di me, non ho avuto il piacere di incontrarla - alla manifestazione ha dichiarato di voler dotare il settore in tempi brevi di una legge sull'enoturismo. Allora sono qui a chiederle di chiarire, perché la norma c'è, c'è, se è suo intendimento rendere pienamente operativa la disciplina a breve. Lo dico perché gli operatori che hanno condiviso con noi quel percorso legislativo

le nostre eccellenze enogastronomiche, oltre ad essere un'enorme risorsa economica per il nostro Paese, rappresentano una straordinaria occasione per promuovere una grande eredità culturale, anche dal punto di vista turistico. In tale contesto, il vino è sicuramente uno dei settori trainanti del nostro *agri-food*, sia a livello nazionale che internazionale, e può essere davvero la forza in più per il nostro Paese. Da qui la necessità di promuovere e valorizzare uno straordinario comparto in crescita che è rappresentato dall'enoturismo. In tale direzione, lo scorso 2 ottobre si è tenuto un incontro con i rappresentanti dell'intera filiera (Coldiretti, Confagricoltura, CIA, Alleanza Cooperative Italiane -Agroalimentare, Unione Italiana Vini, Federvini, Federdoc, Assoenologi) per esaminare il testo di decreto che era stato predisposto, secondo la legge di bilancio 2018, per definire, tra l'altro, le linee guida, i requisiti e gli *standard* minimi di qualità per l'esercizio dell'attività enoturistica. In tale contesto si è convenuto di pervenire ad una soluzione condivisa per una rapida definizione della questione. Al momento siamo in attesa di ricevere le conclusioni cui perverrà la filiera, la cui prossima riunione è fissata per domani, 30 novembre. Mi preme comunque far presente che il nostro intento è quello di garantire la più efficace regolamentazione della fattispecie in esame, con la collaborazione delle Regioni a cui è delegato il turismo, e anche anche dei consorzi. L'obiettivo è dare al sistema Paese delle regole chiare che consentano, in tempi rapidi, di promuovere all'estero l'intero settore del vino, anche attraverso l'incentivazione delle attività connesse all'enoturismo.

che noi apprendiamo con piacere la notizia che ha dato, ma non possiamo dirci soddisfatti, perché di mesi ne sono passati parecchi e la nostra sensazione è che viaggino molto più veloce gli annunci delle cose che si fanno o che si faranno, che non i fatti pratici.

Signor Presidente, signor Ministro, già durante il dibattito sulla Nota di aggiornamento al DEF, noi avevamo sollevato, come Forza Italia, alcune questioni sull'agricoltura. In particolare, abbiamo sottolineato che ormai, sempre più, l'agricoltura non può fare affidamento solo sulla programmazione ma, purtroppo, deve fare i conti con i continui cambi climatici che creano non pochi problemi ai nostri agricoltori. Nel periodo estivo ci sono state forti grandinate fuori stagione, che hanno distrutto gran parte del raccolto. Lo scorso mese, con l'arrivo dell'inverno, si è assistito ad un aumento esponenziale di questi fenomeni, tra l'altro di grande entità, che hanno comportato notevoli danni in tutta Italia. Si parla, come abbiamo potuto vedere anche da stime delle associazioni di categoria, di forti danni

ormai, è un fattore importante con il quale la nostra agricoltura ha a che fare. I danni purtroppo subiti da questo settore sono stimabili in oltre due miliardi di euro, oltre al fondo già previsto, si chiede di sapere se non sia il caso di istituire un fondo particolare per queste calamità climatiche che, nella gran parte dei casi, hanno distrutto la totalità del raccolto

A tal proposito, questo Ministero sta seguendo attentamente e con priorità la situazione di emergenza causata dalle più recenti avverse condizioni meteorologiche che hanno prodotto gravi danni alle infrastrutture, alle vie di comunicazione, alle colture, al patrimonio boschivo, al settore zootecnico nonché alle località turistiche soprattutto costiere. A riguardo, considerata l'estensione del territorio colpito, che ha interessato finora 11 Regioni, e l'importo notevole dei danni causati sia al settore agricolo che al patrimonio forestale, questa Amministrazione si è immediatamente interfacciata con il Dipartimento per la protezione civile e con le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per avviare una rilevazione puntuale dei danni e dei conseguenti fabbisogni per il ripristino delle potenzialità produttive delle imprese agricole e del patrimonio forestale. In tale ambito, questa Amministrazione ha contribuito alla stesura di una prima ordinanza di protezione civile per il settore agricolo che prevede in primo luogo interventi di cui all'articolo 25, comma 2 del decreto legislativo n. 1 del 2018 finalizzati, tra l'altro, a fornire i primi soccorsi al sostegno delle imprese danneggiate dall'evento, per fronteggiare le necessità più urgenti, al finanziamento di interventi per la riduzione del rischio residuo e alla ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture produttive danneggiate. In secondo luogo, si prevede la deroga alle disposizioni del decreto legislativo n. 102 del 2004 per consentire l'attivazione degli interventi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale a fronte dei danni a colture e strutture aziendali assicurabili con polizze agevolate ma non assicurate. In particolare, potranno essere concessi alle imprese agricole: contributi in conto capitale fino all'80 per cento del danno sulla produzione lorda vendibile ordinaria; prestiti ad ammortamento quinquennale per le maggiori esigenze di conduzione aziendale nell'anno in cui si è verificato l'evento e in quello successivo; una proroga delle rate delle operazioni di credito in scadenza nell'anno in cui si è verificato l'evento calamitoso e l'esonero parziale fino al 50 per cento del pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali propri, dei propri dipendenti, contributi in conto capitale per il ripristino delle strutture aziendali danneggiate e per la ricostituzione delle scorte eventualmente compromesse o distrutte. Inoltre, compatibilmente con le esigenze primarie delle aziende agricole, potranno essere adottate anche misure volte al ripristino delle infrastrutture connesse all'attività agricola tra cui quelle irrigue e di bonifica con onere della spesa a carico del Fondo di solidarietà nazionale. La ricognizione dei danni è stata avviata con le Regioni ed è propedeutica anche alla presentazione della richiesta di attivazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea, con il quale sarà possibile integrare finanziariamente la dotazione dell'ordinanza di protezione civile per la realizzazione di alcune attività previste dalla stessa come, ad esempio, il ripristino delle infrastrutture e dei servizi, la realizzazione di strutture di alloggio per soddisfare le necessità immediate anche della popolazione rurale, la ripulitura immediata delle zone danneggiate, comprese le zone naturali. Aggiungo che su iniziativa del Presidente del Consiglio dei ministri, è in fase di ultimazione la ricognizione degli interventi da realizzare con la massima priorità e urgenza al fine di combattere il fenomeno del dissesto idrogeologico e mettere in sicurezza il territorio, attività alla quale questo Ministero ha partecipato attivamente proponendo un piano straordinario di opere da realizzare a cura dei consorzi di bonifica e dei diversi soggetti cui è affidata la gestione delle superfici forestali, volte a ripristinare la funzionalità e l'efficienza idraulica del reticolo idraulico del Paese. In un'ottica di equilibrio strategico delle priorità d'intervento del Governo, finalizzate al rilancio del sistema Paese, tutto il mio impegno - anche in questa delicata sessione di bilancio - è volto a consentire che il comparto agricolo possa essere messo nelle condizioni di superare anche quest'ultima crisi determinata dagli avversi eventi meteorologici che hanno colpito la Nazione.

della sua risposta, anche perché vedremo poi, in questa sessione di bilancio, come evolverà la situazione e quali saranno le misure concrete per andare incontro Tra l'altro, mi permetto di suggerire, qualora fosse possibile, di dare un'indicazione anche alle Regioni, perché molto spesso non riescono a spendere i fondi del piano di sviluppo rurale, per quanto riguarda sia il comparto agricolo, sia quello ambientale, in modo da poter dare un ulteriore contributo alla risoluzione di questi problemi.

Signor Presidente, signori rappresentanti del Governo, mi rivolgo al Ministro dei beni e delle attività culturali. L'area archeologica di Sibari è stata la prima colonia fondata dagli Achei sulla costa ionica della Calabria. Data la protezione naturale costituita dalle foci di due fiumi e la fertilità della pianura in cui venne fondata, a Sud del golfo di Taranto, la colonia in breve tempo divenne ricca e famosa, riconosciuta come la più potente delle città magnogreche, tanto da ricoprire una posizione egemonica su un vastissimo territorio, tale da essere considerata impero sotto il controllo di Sibari. Le profonde modifiche del territorio di Sibari, quali l'avanzamento della linea di costa, dovuto ai depositi fluviali del Crati e del Coscile, e le modifiche degli alvei dei due fiumi avevano nei secoli reso difficile la ricerca archeologica. L'esplorazione scientifica del territorio di Sibari ha avuto inizio nel 1879 e si sono avute importanti scoperte quali la necropoli ellenistica di Turi e la necropoli enotria ed un insediamento del periodo bronzo-ferro all'area di Torre Mordillo. Fin da subito risultò evidente la complessa stratigrafia, dovuta alla sovrapposizione di tre città sullo stesso sito, seppur non totale e con diversa estensione. Negli ultimi vent'anni sono stati stanziati, per il recupero e la valorizzazione del parco archeologico, circa 18 milioni di euro per mettere in sicurezza idrogeologica per mezzo di trincee drenanti, per costruire nuovi edifici per l'accoglienza turistica, per costruire e arredare magazzini e sale del museo e per aprire nuovi scavi archeologici. In particolare, dopo l'alluvione del 2013, sono state messe in opera alcune trincee drenanti, mai usate prima in un sito archeologico, che avrebbero dovuto risolvere in maniera definitiva non solo il problema della risalita di acqua dalla falda, ma anche quello dello smaltimento di acqua piovana e di scorrimento, anche se prima dell'alluvione del 2013 a tenere più o meno all'asciutto le strutture dei monumenti della falda freatica sono stati i *wellpoint*. Le chiedo quali iniziative intenda mettere in atto intenda mettere in atto il Ministero in indirizzo, sia per restituire l'area alla fruibilità del pubblico, che per conoscere come siano stati utilizzati i finanziamenti finora erogati e quali azioni intenda intraprendere per garantire una maggiore tutela, manutenzione e conservazione non solo dell'area archeologica di Sibari, ma del nostro immenso patrimonio archeologico nel suo complesso, compreso quello considerato minore ma ricadente in una Regione con termine a Matera, capitale europea della cultura 2019, visto che l'evento potrebbe essere da volano per lo sviluppo anche dei territori contigui.

e del suo carattere di pregio spiccatamente archeologico, ha assunto carattere perentorio la salvaguardia di ogni singolo manufatto in esso esistente e, conseguentemente, l'integrità dell'intero sito è stata l'obiettivo primario fin qui perseguito e che continueremo naturalmente

tutti i lavori eseguiti sono redatti certificati di regolare esecuzione o verbali di collaudo. Nell'ambito dei fondi PON cultura sono stati da ultimo individuati anche ulteriori 2 milioni di euro, di più IVA già contrattualizzati per lavori di musealizzazione e allestimento. Questi lavori sono ancora in fase di esecuzione. Per quanto riguarda quello che è successo, l'interrogante ha giustamente sottolineato il problema delle trincee drenanti. Fino a due anni fa il

ci eravamo accorti che esse avevano costi di esercizio elevati e, quindi, si era deciso di passare a trincee drenanti, che è la prima volta che vengono utilizzate in un sito archeologico di questo tipo. 3 ottobre le trincee drenanti hanno qualche problema e non riescono più a drenare quanto dovrebbero. Per fortuna, abbiamo sul sito ancora tre pompe drenanti che sono potenzialmente in funzione, quindi per le emergenze abbiamo una capacità di risposta. Sono d'accordo che non bastano per assicurare l'apertura del sito, conseguentemente sono allo studio progetti di fattibilità per, probabilmente, associare a un ripristino delle trincee drenanti una capacità di pompaggio delle acque di faglia per consentire che il sito non venga chiuso, ma sia completamente fruibile.

Confido nel suo lavoro, che vedo proficuo e continuo. La ringrazio e ci impegneremo insieme.

che ha causato la morte di due dipendenti - hanno riportato l'attenzione sulla necessità di garantire la sicurezza all'interno dei luoghi e istituti della cultura e del patrimonio culturale nazionale. Sul tema lei, signor Ministro, è intervenuto in più sedi, affermando l'impegno del Governo per dare priorità alla sicurezza e all'integrità dei luoghi della cultura e dello stesso patrimonio nazionale, al fine di tutelare l'attività dei dipendenti e garantire ai visitatori una fruizione priva di rischi.

importante stanziamento, il Ministero abbia previsto altre misure che vadano nella direzione di un'effettiva attuazione del piano per la messa in sicurezza e la formazione antincendio in tutti i siti italiani, per la salvaguardia dei visitatori, dei lavoratori e delle opere stesse.

Ricordo anch'io molto bene quello che è successo il 20 settembre, perché sono mancati due colleghi, Piero Bruni e Filippo Bagni ed è veramente molto difficile confrontarsi con le famiglie

Lo Stato non ha la stessa attenzione nel chiedere a se stesso quello che chiede, ad esempio, ad un soggetto privato, quindi diversi luoghi della cultura non sono a posto dal punto di vista della sicurezza. Cominciamo a partire da questo. Questa

che ho smobilizzato con un decreto del 25 ottobre per realizzare un piano straordinario pluriennale di sicurezza antincendio, che sarà finanziato interamente dal Ministero. Il piano riguarderà 314 sedi di istituti e luoghi della cultura e ha come obiettivo quello di migliorare sensibilmente la sicurezza dei dipendenti, dei visitatori e del patrimonio culturale. Sono tanti gli interventi relativamente di entità minore, perché quello che abbiamo visto è che, in alcuni casi, magari si erano spesi milioni di euro ristrutturazione, ma mancava quel pezzettino aggiuntivo per fare la scala antincendio in più, il maniglione antipanico in più e quindi per mettere lo Stato in condizioni di rispondere in modo totale alle esigenze di sicurezza. Questo è qualcosa che è successo in passato e il mio impegno è che non accada più in futuro. Per far funzionare questo piano lavoreremo insieme ai Vigili del fuoco,

proposito, tengo a dire che, quando parliamo di formazione dei dipendenti, deve partire dal più alto livello gerarchico all'interno dell'istituzione: se i dirigenti non fanno il corso antincendio, non possono pretendere

creata apposta per occuparsi di questo delicatissimo problema e, più generale, dell'emergenza all'interno del patrimonio, che sarà sotto la direzione del prefetto Fabio Carapezza Guttuso. Il Ministero partecipa inoltre, insieme al Ministero della difesa, al progetto denominato «Duplice uso sistemico» sull'impiego innovativo delle Forze armate al servizio del Paese: si tratta di utilizzare i dati che la Difesa ha a disposizione, attraverso l'uso dei satelliti e dei droni, per monitorare eventuali fenomeni di dissesto idrogeologico legati ai beni

Signor Ministro, sono molto lieta di ascoltare queste sue parole. Mi auguro che questo sia il primo passo per una nuova stagione all'interno del Ministero, dedicata a un grande piano di manutenzione ordinaria, perché, come ci siamo già detti in altre occasioni, il mondo dei beni culturali ha bisogno di un piano di manutenzione ordinaria. Manca l'ordinario, non è mai stato fatto e nella Legislatura precedente ci si è molto dedicati alle operazioni di grande effetto mediatico e non si è prestata cura, invece, a quella che dovrebbe essere la prima preoccupazione, ovvero quella di salvaguardare i nostri luoghi, quotidianamente. Mi auguro che con il prossimo anno si inauguri questa stagione nel Ministero, si possa mettere a punto un grande piano di manutenzione e che poi, magari nella manovra finanziaria dell'anno venturo, possano essere destinate le risorse

Comunico che il Presidente del Senato e il Presidente della Camera dei deputati hanno proceduto alla nomina dei componenti della Commissione parlamentare di vigilanza sull'anagrafe tributaria.

sono convocate, per la loro costituzione, mercoledì 5 dicembre, nella sede di Palazzo San Macuto, in via del Seminario, secondo gli orari di seguito indicati: ore 8,30, Commissione parlamentare per la semplificazione e Commissione parlamentare di vigilanza sull'anagrafe tributaria; ore 14,00, Commissione parlamentare per le questioni regionali e Commissione parlamentare di controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale.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

Signor Presidente, gentili colleghe e colleghi, in vista del *derby* calcistico di serie B tra Crotone e Cosenza di lunedì 26 novembre, la rubrica del TGR Calabria «Buongiorno Regione» ha ospitato Giancarlo Ciabattari, un ex calciatore che negli anni Sessanta e Settata giocò per la squadra bruzia, ma fu anche prestato ai cugini pitagorici. Oltre che in qualità di vecchia gloria di entrambe le squadre, Ciabattari è stato presentato come autore di due libri, i cui proventi saranno destinati in beneficenza. Gli spettatori sono però rimasti allibiti nel sentire che il primo romanzo, del 2012 e ripubblicato l'anno scorso, s'intitola «Zio Luigi, l'ultimo uomo d'onore».

lettori. Sui siti *on line* dov'è possibile acquistarlo, infatti, la moglie del Ciabattari, calabrese, si esprime come segue: «Nel racconto del libro "Zio Luigi. L'ultimo uomo d'onore"

o addirittura mitizzare esponenti della criminalità organizzata. Per di più, il rapporto malato mafia-calcio si alimenta da sempre di una certa qual tolleranza nei confronti di individui e situazioni la cui valenza può eventualmente sfuggire all'uomo comune, ma non può né deve sfuggire agli organi di informazione. Concludo, signor Presidente, dicendo che mi riprometto d'investire del caso la Commissione di vigilanza Rai e che ho già presentato un esposto all'ordine dei giornalisti e alla Federazione nazionale della stampa italiana, sperando che in futuro tutti i professionisti della comunicazione prestino maggiore attenzione a temi così delicati per il nostro Paese.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, intervengo in Aula per portare all'attenzione dell'Assemblea una vicenda incresciosa che vede, ancora una volta, coinvolta la mia terra, la Calabria. Alcuni giorni or sono, è andato in onda il *reportage* di un programma televisivo che ha messo in luce alcune anomalie riguardanti lo svolgimento di una procedura di selezione pubblica per autisti delle Ferrovie della Calabria, società di proprietà della Regione. In sede di prova, agli aspiranti autisti sarebbero stati forniti, come del resto è prassi, un cedolino con i dati anagrafici prestampati, un foglio con le domande e uno per le risposte, da indicare annerendo le apposite caselle. Ebbene, sul cedolino e sul foglio delle risposte vi erano appositi spazi nei quali applicare una coppia di codici a barre adesivi. È evidente come tale meccanismo, ideato per associare, anonimamente, il compito al concorrente, non abbia però i requisiti per garantire la paternità dell'elaborato, diversamente da quanto previsto in diverse procedure concorsuali di altre Regioni d'Italia, dove il codice a barre del cedolino dev'essere controfirmato.

in misura trascurabile. Ulteriori dubbi sul bando sono emersi su alcune testate giornalistiche locali, nelle quali è stato ampiamente messo in risalto il fatto che la data originariamente prevista per lo svolgimento della prova preselettiva sia stata rinviata per permettere ad alcuni candidati

emerso dagli organi di stampa sulla correttezza dello svolgimento del concorso e venga fatta luce il prima possibile sui fatti sopra descritti, che, se corrispondessero a quanto esposto, recherebbero grave nocumento alle legittime richieste di giustizia e trasparenza,